per ritornare su un aspetto che abbiamo ieri denunciato e cioè quello del baratto tra le forze politiche di maggioranza. Io spero che i colleghi della maggioranza…

Sì, tutte le bandiere vanno rispettate, soprattutto il Tricolore. Soprattutto il Tricolore va rispettato

Signora Presidente, lo dico perché aver costretto il Parlamento ad una seduta notturna che è finita questa mattina alle 7,50 dà la dimostrazione plastica del baratto avvenuto che abbiamo denunciato per mesi. *(Applausi)*. L'Aula di Montecitorio è stata costretta questa notte a votare, emendamento dopo emendamento, quando non c'era alcuna urgenza. Presidente Malan, non c'era alcuna urgenza. Lo dico per noi, perché poi dobbiamo definire le modalità con le quali convivere in queste Aule. Quello che è avvenuto a Montecitorio è grave, lo denunciamo e ribadiamo che il baratto fa solo male al Paese. Non ci lasciate altro scampo che la raccolta firme per un *referendum* che boccerà lo "spacca Italia" di Calderoli, perché finirà così. una cosa che però ci preoccupa di più. Signora Presidente, lo dico qui e poi con i colleghi Presidenti dei Gruppi di opposizione sono sicuro che riusciremo a coordinare l'azione. Signora Presidente, io le chiedo sin da ora di chiedere al Governo di non prestarsi alla firma di alcuna pre-intesa con nessuna Regione fino a quando il ministro Giorgetti non ci avrà detto dove sono le risorse, quando i due rami del Parlamento delibereranno per il finanziamento dei LEP e, soprattutto, quando saranno definiti i livelli essenziali delle prestazioni. Sul trasporto pubblico locale, sull'assistenza, dagli asili nido agli anziani, sulla sanità e sulla scuola non si fa propaganda politica. *(Applausi)*. Avete fatto tanta propaganda politica, ma quella è la vita vera degli italiani. Quindi, signora Presidente, il baratto c'è stato ed è andato in onda, purtroppo, questa notte. All'alba, gli italiani si sono svegliati ritrovandosi con lo "spacca Italia" che è diventato legge. Noi chiediamo, innanzi tutto, alla Presidenza la convocazione della Conferenza dei Capigruppo che era già programmata, ma mancava l'orario. Mi auguro che si

Aula il ministro Giorgetti che dovrà spiegarci come intendono andare avanti, visto che la legge sull'autonomia, lo "spacca Italia" di Calderoli, è in vigore, ma non c'è un euro, perché dentro la legge stessa avete

Il punto non è che questi due provvedimenti erano entrambi nell'agenda di Governo dei due principali partiti del centrodestra. Lo sappiamo perfettamente. Lo abbiamo letto il programma di Governo i cittadini l'hanno votato. Quindi, sappiamo bene che l'autonomia differenziata e il presidenzialismo (perché all'epoca c'era il presidenzialismo nel programma di Fratelli d'Italia) erano contenuti all'interno del programma di Governo con cui le forze di destra si sono presentate alle elezioni. Il punto che devono spiegare agli italiani è come conciliano questi due provvedimenti, che sembrano ispirati a logiche completamente opposte. Su questo non hanno saputo dire niente in tutti questi mesi. *(Applausi)*. Quelli che hanno sostenuto, in tutti questi anni, addirittura che la riforma del Titolo V fosse sbagliata,

al pensiero dei loro padri fondatori, ma questo è un problema loro, naturalmente, non un problema mio. Ora riconoscono l'autonomia differenziata, che dovrebbe essere quanto di più distante da quel tipo di cultura politica Il punto non è che tali riforme erano entrambe contenute nel programma di Governo. Il punto è che parliamo di due provvedimenti totalmente in contraddizione l'uno con l'altro, che hanno solo una cosa in comune, come abbiamo detto in tutti questi mesi,

avremmo un Paese in cui c'è un Primo Ministro che accentra tutti i poteri; quali sono questi poteri, però, non è troppo chiaro, perché nel frattempo se ne decentra una parte rilevantissima ai Presidenti di Regione, anzi ai governatori, perché a quel punto saranno davvero governatori. Governeranno le Regioni come se fossero dei piccoli Stati e voi capite bene che il combinato disposto di questi due provvedimenti crea

come si tengono assieme questi due principi che sono culturalmente radicalmente diversi? Io penso che su questo, in tutti questi mesi,

per quale motivo questo scambio deve rimanere a due, perché devono esserci soltanto premierato e autonomia differenziata? Aggiungiamo anche la riforma della giustizia nello scambio, così lo facciamo perfettamente e ci accontentiamo tutti. Questo è ciò che sta accadendo plasticamente sotto gli occhi del Paese. Capite bene che, dal nostro punto di vista, a questa logica abbiamo il diritto o anzi, io penso, addirittura il dovere di mettere in campo l'opposizione più forte possibile. In Parlamento naturalmente i numeri li avete perché siamo stati sufficientemente stolti qualche mese fa, stolti qualche mese fa, ma questa cosa certamente non accadrà più nel futuro prossimo e, soprattutto, quando la parola spetterà ai cittadini, vedrete che queste pagine tristi che abbiamo vissuto,

che sarà più o meno sulla stessa lunghezza d'onda, perché sono la dimostrazione plastica di quanto state rosicando.

noi vorremmo portare un ulteriore elemento di riflessione a supporto dell'istanza, che condividiamo, avanzata dal presidente Boccia di richiedere una immediata audizione Signora Presidente, colleghi, oggi l'Italia è entrata nella procedura di infrazione. avrebbe detto che la ricreazione è finita. Mentre noi siamo stati immersi dentro i fuochi fatui di una campagna elettorale giocata all'insegna degli effetti speciali,

e i conti pubblici del nostro Paese non sono in ordine, non sono in linea, non sono adeguati. Questa è la drammatica verità. Visto che si discute di autonomia differenziata che deve essere finanziata, sarebbe davvero interessante comprendere come questo possa avvenire nella misura in cui il meccanismo che contempla la procedura di infrazione contiene l'obbligo per il Governo di presentare un piano fiscale e strutturale di riordino della spesa pubblica nel nostro Paese che preveda riforme a medio termine, che preveda tagli di spesa e che possa prevedere, nel caso in cui i tagli di spesa non vengano realizzati, incrementi di tasse. Questo perché mentre voi salite sui palchi dei comizi a raccontare che arriverà l'autonomia differenziata e che quindi, improvvisamente, saremo tutti più ricchi, bisogna trovare tra i 10 e i 12 miliardi per rispettare le regole dell'Unione europea, che prevedono nel Patto di stabilità - che voi avete definito all'interno del Consiglio europeo, signori della maggioranza, signori del Governo, non lo hanno fatto i i poteri forti, Soros o qualche altro globalista che voleva realizzare chissà quale macchinazione, ma l'avete concordato, definito e sottoscritto voi - l'obbligo di ridurre di mezzo punto percentuale l'anno il *deficit* strutturale. Ci volete spiegare per favore come lo volete fare, visto che i 10 miliardi che avete stanziato per il taglio del cuneo fiscale a debito

il nostro Paese torni a ballare, una situazione che noi vogliamo assolutamente evitare. Mentre siamo immersi in una situazione da fumeria d'oppio, nella quale discutiamo di cose irreali, la realtà si sta imponendo, con tutte le sue conseguenze. Pertanto, anche noi siamo dell'opinione che debba essere convocata la Conferenza dei Capigruppo e che debba essere immediatamente calendarizzata un'audizione del ministro Giorgetti, perché tutti questi aspetti rientrano anche nella responsabilità di un Governo che si è presentato in quest'Aula con un DEF senza avere in alcun modo detto come tutti questi aspetti sarebbero stati affrontati. Adesso l'imbuto si è ristretto e, cari signori, ci dovete dire come pensate di farci passare da quel pertugio.

per i successi degli altri, un po' preoccupati se quei successi rappresentano un fallimento per il Paese, questo ovviamente sì. *(Applausi)*. Aggiungo molto poco a quanto detto dai miei colleghi, che condivido; dico soltanto che qualche volta il destino, il fato

che parla della lungimiranza e dell'intuizione dei Padri costituenti: quella Costituzione che, con l'autonomia differenziata fatta in un modo scellerato e con il premierato voi state distruggendo, è oggi sui testi dei maturandi che vorranno analizzarla e diranno la loro su quanto sia fondamentale difenderla. *(Applausi)*. Questo è sufficiente. Penso che siano altri a dover rosicare oggi.

Il cambiamento climatico è stato trascurato in questo accenno di seduta. I problemi sono molteplici: gli Houthi che bombardano le navi nel Mar Rosso, Gaza (e lo dico con serietà), l'attacco all'Ucraina. I problemi dell'umanità - ripeto - sono molteplici, quindi è bene che il Parlamento la mattina li ricordi. Non ho capito quindi di che cosa stiamo parlando. Mentre entravo in Aula ho sentito commenti sulla seduta della Camera

chi lo può usare e come. Quanto agli incidenti parlamentari, mi sembra il "processo del mercoledì". Vi ricorderete che andava in onda «Il processo del lunedì», con il compianto Aldo Biscardi. Stiamo facendo il dibattito del giorno dopo al bar: legge mi piace, quella non mi piace; spiegateci il programma; non si abbina la cravatta con il vestito e il premierato con l'autonomia regionale. È un dibattito sull'universo mondo, ma non mi scandalizza, perché il Parlamento è fatto per parlare e per confrontarsi. Sapevo però che all'ordine del giorno c'era un provvedimento urgentissimo sulla cybersicurezza: era urgentissimo quando doveva essere utilizzato per posporre il voto sul premierato; adesso è meno urgente. Ci manca solo il VAR

altri organismi parlamentari per decidere anche come si usano i fondi dei Gruppi parlamentari della Camera e del Senato, visto che giustamente qui si parla di tutto. Siamo al processo del mercoledì, quindi anch'io voglio il moviolone sugli argomenti che chiedo io.

ho dato a ciascun Gruppo la possibilità di esprimersi. Adesso attendo ovviamente anche l'intervento del presidente Malan per comprendere cosa riportare al presidente La Russa.

presidente Gasparri, inclusa la citazione di Antonio Gramsci con la quale ha esordito. Io voglio fare un'altra citazione. Un collega che è stato senatore per parecchie legislature, che è stato Capo dello Stato ed anche Presidente del Senato, diceva che non bisognerebbe neppure menzionare l'altro ramo del Parlamento, tutt'al più denominandolo in questo modo. Diceva inoltre che bisogna fare come a Oxford e Cambridge, dove, parlando ciascuno dell'altra università, la definiscono semplicemente *the other place*, l'altro posto. Non so se lui avesse ragione, anche perché il presidente Cossiga ha sperimentato sulla sua pelle che il sacrale rispetto per il Capo dello Stato nel suo caso fu dimenticato. *(Applausi)*. Ripeto, il sacrale rispetto del Capo dello Stato nel suo caso fu dimenticato, con insulti pesantissimi anche nelle Aule parlamentari - peraltro spesso adeguatamente ricambiati - e anche con l'avvio della messa in stato d'accusa. Ebbene, non penso che l'apertura di seduta per discutere di quanto avviene nell'altro ramo del Parlamento. Detto questo, ovviamente ciascuno usa la facoltà di parola come crede. Riguardo all'unica richiesta sull'ordine dei lavori e la Conferenza dei Capigruppo, ci rimettiamo

finestra"). A conclusione di questo giro di interventi, ovviamente senza alcun commento da parte mia, come è fin troppo ovvio che debba essere, ma solo per il verbale, il presidente Boccia ha fatto menzione non tanto

dalla Camera. Il testo del provvedimento si compone di 24 articoli, suddivisi in due Capi. Nell'illustrare il contenuto del disegno di legge, si soffermerà sulle parti di interesse della 1a Commissione, ovvero sugli articoli da 1 a 15, ricompresi nel Capo I, lasciando quindi la parola al relatore della 2a Commissione per l'illustrazione dei restanti articoli. L'articolo 1 è volto a prevedere un più ampio obbligo di notifica di incidenti rilevanti per la cybersicurezza per soggetti ulteriori rispetto a quelli già ricompresi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica istituito dal decreto-legge n. 82 del 2021. Il comma 2 indica le modalità con le quali effettuare la notifica. Il comma 3 dispone che gli obblighi di notifica si applichino per alcuni soggetti a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. In base al comma 4, i soggetti indicati al comma 1 possono anche effettuare notifiche volontarie di incidenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di notifica. I commi 5 e 6 attengono alle sanzioni per la violazione dell'obbligo di notifica, mentre il comma 7 esclude alcuni L'articolo 2 prevede che le amministrazioni e gli enti pubblici e altri soggetti che forniscono servizi pubblici, qualora siano oggetto di segnalazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale circa specifiche vulnerabilità cui essi risultano potenzialmente esposti, debbano provvedere tempestivamente, e comunque non oltre quindici giorni dalla comunicazione, all'adozione degli interventi risolutivi indicati dalla stessa Agenzia. L'articolo 3 stabilisce che i soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica provvedano, oltre che alla notifica, anche alla segnalazione degli incidenti che intervengono su reti, sistemi informativi e servizi informatici di loro pertinenza L'articolo 4, introdotto dalla Camera, prevede che i dati relativi a incidenti informatici siano raccolti, sulla base degli adempimenti di notifica previsti a legislazione vigente, dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che ne cura la pubblicità come dati ufficiali di riferimento degli attacchi informatici. L'articolo 5 prevede la possibilità di far partecipare alle riunioni del Nucleo per la cybersicurezza ulteriori soggetti, tra i quali rappresentanti della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e rappresentanti della Banca d'Italia, consente al Presidente del Consiglio dei ministri di disporre il differimento degli obblighi informativi e delle attività di resilienza in capo all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nei casi in cui questo sia considerato strettamente necessario dai servizi di sicurezza della Repubblica. L'articolo 7, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, modifica la composizione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), disponendo che del Comitato facciano parte anche il Ministro dell'agricoltura, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'università e della ricerca. L'articolo 8 istituisce, per le pubbliche amministrazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, ove non sia già presente, la struttura preposta alle attività di cybersicurezza, L'articolo 9, introdotto dalla Camera, attribuisce alle strutture preposte alle attività di cybersicurezza nelle pubbliche amministrazioni la funzione di verificare che i programmi e le applicazioni informatiche e di comunicazione elettronica rispettino le linee guida sulla crittografia, nonché quelle e che non contengano vulnerabilità note. L'articolo 10, interamente sostituito nel corso dell'esame alla Camera, modifica il decreto-legge n. 82 del 2021, al fine di valorizzare l'utilizzo della crittografia quale strumento di difesa cibernetica e istituisce il Centro nazionale di crittografia presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. L'articolo 11 definisce termini e modalità per l'adozione del regolamento che stabilisce i criteri, anche temporali, per l'accertamento, la contestazione e la notificazione delle violazioni della normativa in materia di cybersicurezza e l'irrogazione delle relative sanzioni di competenza dell'Agenzia. del decreto-legge n. 82 del 2021, stabilisce che i dipendenti appartenenti al ruolo del personale dell'Agenzia che abbiano partecipato, nell'interesse e a spese dell'Agenzia stessa, a specifici percorsi formativi di specializzazione, per i due anni successivi alla data di completamento dell'ultimo dei predetti percorsi formativi non possano essere assunti, né assumere incarichi, presso soggetti privati per svolgere mansioni in materia di cybersicurezza.

L'articolo 15, aggiunto dalla Camera, introduce nel testo dell'articolo 16 della legge di delegazione europea 2022-2023 nuovi principi e criteri direttivi specifici a cui il Governo dovrà attenersi nel recepimento della normativa europea in materia di resilienza operativa digitale per il settore finanziario.

rilevante in crescita esponenziale. Gli attacchi cibernetici sono sempre più frequenti e creano non solo insicurezza per i nostri sistemi, ma anche la possibile divulgazione di dati sensibili. Tra tutti voglio fare solo un riferimento a quelli in materia sanitaria: ormai non c'è Regione, non c'è Provincia, non c'è USL o ASL che non sia stata colpita da questi attacchi che non provocano solo la sottrazione di dati sensibili, ma creano anche danno all'erogazione dei servizi ai cittadini, perché, ogniqualvolta si verificano, ci sono periodi di interruzione nella prenotazione delle visite. Sappiamo quanto sia rilevante la necessità di accelerare visite e prestazioni per le nostre comunità in tema sanitario. Quindi, è particolarmente importante che questo provvedimento sia stato approvato rapidamente alla Camera, col contributo

non servirà a impedire qualsiasi attacco cibernetico ma, sulla base dell'esperienza passata, dà degli strumenti aggiuntivi alle pubbliche amministrazioni per cercare di prevenirli, evitarli e segnalarli con tempismo per limitare i danni nel maggior modo possibile. Quindi, ringrazio tutti i componenti delle Commissioni per il lavoro svolto e consegno il testo integrale del mio intervento

L'articolo 16 reca modifiche al codice penale in materia di prevenzione e contrasto dei reati informatici. Occorre sottolineare preliminarmente che le disposizioni recate dal comma 1, lettera *a)*, risultano conseguenti alle modifiche introdotte dalla lettera dello stesso comma 1, del quale si dirà in seguito. Il comma 1, lettera *b)*, modifica poi l'articolo 615-*ter* del codice penale (accesso abusivo a un sistema informatico telematico), ampliandone l'ambito di applicazione della fattispecie e inasprendo il trattamento sanzionatorio. Il comma 1, lettera *c)*, modifica l'articolo 615-*quater* del codice penale e la disposizione, oltre a modificare la definizione della fattispecie delittuosa, ampliando il dolo specifico previsto per la configurabilità della fattispecie attraverso la sostituzione della nozione di profitto prevista dal testo vigente con quella più ampia di vantaggio, ne ridefinisce anche le aggravanti. La lettera *d)* del comma 1 abroga l'articolo 615-*quinquies* del codice penale, il cui contenuto è però integralmente riprodotto nel nuovo articolo 635-*quater*. Il comma 1, lettera *e)*, interviene sull'articolo 617-*bis* del codice penale prevedendo una circostanza aggravante che ricorre nel caso di commissione del fatto da parte di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri da un investigatore privato anche abusivo o con abuso della qualità di operatore di sistema. Il comma 1, lettera *f)*, interviene sull'articolo 617-*quater* modificandone in particolare le circostanze aggravanti. Il comma 1, lettera *g)*, modifica l'articolo 617-*quinquies* del codice penale, intervenendo anche in questo caso sulle aggravanti. Il comma 1, lettera *b)*, apporta modifiche all'articolo 617-*sexies*, prevedendo l'innalzamento della pena per la fattispecie aggravata. Il comma 1, lettera *i)*, reca una disposizione di coordinamento volta a modificare la rubrica del capo III-*bis* del titolo XII del libro secondo del codice penale, ora denominata «Disposizioni comuni», conseguentemente all'introduzione dell'articolo 623-*quater*. Il comma 1, lettera *l)*, prevede l'inserimento nel codice penale dell'articolo 624-*quater* in materia di circostanze attenuanti per i delitti di cui agli articoli 615-*ter* (accesso abusivo a un sistema informatico telematico), 615-*quater*, 617-*quater*, 617-*quinquies* e 617-*sexies*. Il comma 1, lettera *m)*, aggiunge un comma all'articolo 629 del codice penale (estorsione) che punisce con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000 la fattispecie del delitto di estorsione mediante reati informatici realizzata dalla costrizione di taluno a fare o omettere qualcosa, procurando a sé o altro ingiustificato profitto mediante condotte o la minaccia di compierle. Si prevedono inoltre la reclusione da otto a ventidue anni e la multa da euro 6.000 a euro 18.000 se ricorre taluna delle circostanze aggravanti del delitto di rapina. Il comma 1, lettera *n)*, interviene sull'articolo 635-*bis* prevedendo l'innalzamento della pena per la fattispecie semplice, modificando la disciplina della fattispecie aggravata. Il comma 1, lettera *o)*, modifica l'articolo 635-*ter* intervenendo sulla definizione della fattispecie delittuosa e apportando modifiche alle circostanze aggravanti. Il comma 1, lettera *p)*, interviene sull'articolo 635-*quater* prevedendo un innalzamento della pena per la fattispecie semplice e l'ampliamento della fattispecie aggravata riguardo al danneggiamento di sistemi informatici o telematici. Il comma 1, lettera *q)*, introduce nel codice penale l'articolo 635-*quater*.1 (detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico). Il primo comma del nuovo articolo riproduce il vigente articolo 615-*quinquies*

o telematico) -* Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la disciplina il reato di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse. Rispetto alla fattispecie vigente, si prevedono un innalzamento sanzionatorio e la sostituzione della nozione di servizi informatici o telematici di pubblica utilità con quella di servizi informatici o telematici di pubblico interesse. Il comma 1, lettera *s)*, prevede l'inserimento nel codice penale dell'articolo 639-*ter* in materia di circostanze attenuanti per i delitti di cui all'articolo del codice penale 629, terzo comma, introdotto dalla lettera Attraverso una modifica approvata nel corso dell'esame presso la Camera sono state aggiunte tre ulteriori lettere al comma 1. L'intervento principale è quello contenuto alla lettera *t)*, che inserisce all'articolo 640 del codice penale, secondo comma, una nuova circostanza aggravante del reato di truffa, nel caso in cui il fatto sia commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui individuazione. La medesima lettera *t)*, inoltre, prevede l'applicazione della nuova circostanza aggravante del reato di truffa al regime di procedibilità a querela della persona offesa. Passando all'articolo 17, esso reca modifiche al codice di procedura penale finalizzate a recepire gli interventi in materia di prevenzione e contrasto dei reati informatici introdotte dall'articolo 16. La lettera *a)* interviene sull'articolo 51 del codice di procedura penale, che al comma 3-*quinquies* reca il catalogo dei reati informatici attribuiti alla competenza del procuratore distrettuale. Oltre a sopprimere il riferimento all'abrogando articolo 615-*quinquies*, sono inseriti i riferimenti all'articolo 635-*quater*.1 e 635-*quinquies* del codice penale, nonché al delitto relativo alla comunicazione di dati, informazioni o elementi di fatto falsi tesa a ostacolare o condizionare la formazione e trasmissione dell'elenco di reti, sistemi informatici e informativi da parte degli operatori compresi nel perimetro di sicurezza cibernetica, le procedure di affidamento delle forniture di strumenti destinati ai servizi e ai sistemi informatici o le attività ispettive e di vigilanza sui reati contro i sistemi informatici e i servizi informatici. L'articolo 18 reca poi alcune modifiche alle norme sui collaboratori di giustizia, di cui al decreto-legge n. 8 del 1991. La lettera *a)* estende le condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione per i collaboratori di giustizia anche nei confronti degli autori di gravi delitti informatici, in relazione ai quali al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sono riconosciute funzioni di impulso nei confronti dei procuratori La lettera *b)* estende anche per i reati informatici la comunicazione al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo della proposta di ammissione alle speciali misure di protezione in favore del collaboratore di giustizia. L'articolo 19 estende la disciplina delle intercettazioni previste per i fatti di criminalità organizzata ai reati informatici rimessi al coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. L'articolo 20 interviene sul catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. L'articolo 21 modifica il procedimento di applicazione delle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia e per gli altri protetti, prevedendo che la Commissione centrale debba chiedere il parere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sulla proposta di ammissione alle speciali misure. L'articolo 22 disciplina il rapporto tra l'Agenzia di cybersicurezza nazionale, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, la polizia giudiziaria e il pubblico ministero. L'articolo 23, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede alcune modifiche all'articolo 7 della legge n. 1311 del 1962, recante l'organizzazione e il funzionamento dell'ispettorato generale presso il Ministero della giustizia. L'articolo 24 è di invarianza finanziaria.

il testo che ci accingiamo a discutere e poi a votare è sempre espressione di questo approccio che il Governo reitera ormai da quasi due anni su tutti i problemi di cui intende occuparsi. Anche stavolta non ci siamo discostati dal vecchio schema, che sintetizzerei in un reprimere e condannare; poi, per il resto, il Governo poco altro fa.

di cui ormai ogni cittadino dispone e che sono diffusissimi, contengono una mole di informazioni personali, di dati sensibili, di dati sanitari, di dati economici, di dati che ci profilano, ci profilano, ci caratterizzano e consentono a chi vi ha accesso di conoscere qualsiasi cosa voglia sapere di noi; essi sono talmente tanti da rendere necessaria una strategia di difesa quanto più estesa possibile. Questo, almeno nelle intenzioni generali, è l'intendimento di questo decreto-legge. Pensate che si stima che nel 2025 ci saranno 41 miliardi di *digital device*, cioè di strumenti informatici collegati in rete che condivideranno fra di loro e scambieranno informazioni.

si è sempre battuta per l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza. Ci siamo battuti per la sua istituzione, ci siamo adoperati per rafforzarla, darle operatività e capacità di intervento. in tal senso da questo decreto-legge che alle dichiarazioni sostanziali e programmatiche, alle buone intenzioni, si aggiungesse la sostanza. che si dessero le risorse economiche per far funzionare meglio l'Agenzia nazionale della cybersicurezza e, soprattutto, per mettere in condizione tutti gli altri soggetti che il provvedimento individua come soggetti attivi (cioè come soggetti che sono onerati dell'obbligo di comunicazione, notificazione e denuncia di minaccia o di attacco informatico) di poterlo fare. Ricordiamo che questi soggetti sono le Regioni, le Amministrazioni centrali, le Città metropolitane, le città con oltre 100.000 abitanti, le aziende di trasporto pubblico che abbiano una utenza superiore ai 100.000 abitanti,

cybersicurezza, individuare, anche a loro carico, l'obbligo di comunicazione, di notificazione e denuncia di un attacco informatico

eseguire e soprattutto verificare che la società o che l'ente al quale appartiene e per il quale opera si sia dotato di strumenti di resilienza, di resistenza e di controllo del trattamento dei dati, al fine di evitare e scongiurare l'attacco, adoperandosi immediatamente a dare seguito a tutte le misure necessarie a difendere i dati anche sulle sollecitazioni inviate dall'Agenzia nazionale.

L'approccio che il Governo mantiene nei confronti degli enti locali, delle Regioni e dei rapporti istituzionali si conferma deteriore, accentra

rafforzamento delle misure di contrasto agli attacchi informatici, ha una finalità che forse non è stata chiaramente indicata. Ho ascoltato con attenzione la relazione dei due colleghi senatori

sul codice degli appalti, prevedendo che quando le amministrazioni fanno le gare per dotarsi degli strumenti per il contrasto agli attacchi informatici e, quindi, dispositivi tecnologici, consulenze o servizi che devono implementare all'interno della loro amministrazione, dovranno tener conto di altri parametri, oltre a quelli già previsti nel codice degli appalti. Questi altri parametri constano sostanzialmente di un pacchetto di norme che storicamente potremmo definire protezionistiche. Infatti, si dice

quelle che operano nella comunità europea o quelle che, comunque, hanno un profilo per il quale bisogna preferirle agli altri operatori. Questo ci pone, evidentemente, di fronte a una riflessione. Una normativa del genere si pone in contrasto con l'Unione europea. È ovvio: non ci possono essere norme protezionistiche. Questo il Governo lo sa, ma, purtroppo, si ostina a andare contro le norme generali comunitarie. Quella sulla libera concorrenza è proprio quella che, fra tutte, come principio a questo Governo non piace. È proprio un principio che non sopporta. Non può proprio sentirlo discutere. stiamo ancora aspettando che si risolva il problema delle concessioni balneari. Vedremo se dovremo incorrere ancora in un richiamo da parte dell'Unione europea. *(Applausi)*. che è ancora più interessante e sulla quale entrambi i relatori hanno completamente sorvolato, è quella relativa al divieto, per il personale che ha lavorato all'interno dell'Agenzia nazionale della sicurezza o negli organismi della sicurezza nazionale, di potere, al termine dei percorsi formativi per i quali ha svolto la propria attività al servizio dell'Agenzia o degli altri organismi, organismi, di lavorare liberamente. Quindi, immaginiamo un professionista che partecipa a un corso di formazione all'interno dell'Agenzia nazionale, si specializza e lavora per un certo periodo di tempo all'Agenzia nazionale. Poi questo incarico cessa,

Bastava tutelare la riservatezza con un patto di segretezza, come si fa in tutte le amministrazioni dove si trattano argomenti del genere e materie così delicate. Porre un divieto assoluto e generalizzato significa,

strana! Quello stesso soggetto che, se magari è un collaboratore esterno, per tre anni non potrà più lavorare con nessuno, se invece è un dipendente in servizio che va in pensione, non avrà più alcun vincolo.

del collaboratore di giustizia dei reati informatici. Chi, dopo aver commesso il reato, si adopera con lo Stato per rimediare al reato e alle sue conseguenze, può avere un beneficio pari pari ad uno sconto di pena tra la metà e i due terzi della pena prevista per il reato commesso. Peccato che, nella fretta,

al baratto o, per meglio dire, allo scambio, anzi al mercimonio dei provvedimenti, entrando in una logica spartitoria in virtù della quale i partiti al Governo ne hanno imposto l'esame nell'agenda politica. Sappiamo bene, come abbiamo detto più volte in quest'Aula, che consiste nel premierato a Giorgia, spacca Italia alla Lega Nord e separazione delle carriere dei magistrati a Forza Italia. Si sperava di aver raggiunto il fondo, ma purtroppo al peggio non vi è mai fine. In preda all'euforia di Tele Meloni, seguendo una regola cara ai noti imbonitori televisivi, ormai l'agenda politica è segnata dalle scadenze, siano esse stesse elettorali ovvero legate ad impegni istituzionali. Infatti, la reale ragione della compressione dei tempi di esame del provvedimento ad oggetto dei lavori di questa Assemblea era una disperata corsa al G7, che però non ha raggiunto il suo obiettivo, perché la questione del premierato ha avuto la precedenza in quest'Aula. il tentativo di sbandierare davanti ai *leader* riuniti il fatto che, grazie al Governo Meloni, l'Italia rappresenterà l'avanguardia mondiale in materia di cybersicurezza non è riuscito come avreste voluto. però, come stanno realmente le cose: l'Italia, purtroppo, signor Presidente, si colloca all'ultimo posto dei Paesi del G7 per quanto riguarda il rapporto tra le spese per la cybersicurezza ed il PIL con lo 0,12 Sarei proprio curiosa di sapere se questo sia stato detto dalla presidente del Consiglio Meloni in quel di Fasano. La cybersicurezza è essenziale per garantire un corretto sviluppo economico del Paese; il tessuto connettivo del nostro sistema economico è formato dalle attività delle piccole e medie imprese, ma troppo spesso sono proprio loro i destinatari degli attacchi. La esfiltrazione dei dati personali dei clienti a scopo estorsivo è aumentata del 27 per cento rispetto all'anno scorso. Si dirà che il disegno di legge in oggetto ha novellato l'articolo 629 del codice penale, creando la fattispecie dell'estorsione mediante i reati informatici, ma ciò non è sufficiente. Nella quasi totalità dei casi, infatti, le aziende preferiscono silenziare il cyberfurto accettando l'estorsione, piuttosto che rendere nota l'aggressione *hacker* col rischio del danno reputazionale: preferiscono, insomma, pagare il riscatto e finire nella *black list* dei soggetti pagatori che periodicamente subiscono incursioni. Per capire il fenomeno, occorre stimare le cifre: nel 2022 tale *business* illecito ha toccato cifre altissime in termini di riscatti e proprio a tal fine sarebbe stata utile la diffusione della conoscenza dei temi di cybersicurezza presso le PMI, PMI, al fine di promuovere comportamenti positivi volti al contrasto di tali condotte. Si potrebbe dire, in via in generale, che il Paese tutto necessita di una cultura della cybersicurezza, al fine di rendere consapevoli tutti gli attori in gioco dell'importanza dei temi di cui si tratta. Le modalità attraverso le quali il Governo ha inteso intervenire sulla materia sono indicative di come semplicisticamente si intenda affrontare questi problemi. di dirlo, signora Presidente - aggravio sanzionatorio compiuto, inteso sia come creazione di fattispecie di reato *ad hoc,* sia di aggravanti ad effetto speciale, sia di inasprimento delle sanzioni assistenti, appare infatti totalmente insufficiente ai fini di una compiuta analisi della fattispecie. Non vi è chi non veda, infatti, che la scelta di agire esclusivamente sulla pena per talune ipotesi di reato renderebbe la stessa disallineata rispetto al principio di proporzionalità della stessa, andando ad annullare l'effetto deterrente della sanzione, poiché il reo avrà l'impressione di soffrire di una pena ingiusta, in quanto scollata rispetto al principio di offensività della condotta. In più,

nulla dice o consiglia in merito alla necessità di adeguare la legislazione interna degli Stati in ordine all'impianto repressivo penale mediante l'introduzione di nuove fattispecie di reato o di aggravanti speciali, con relativo meccanismo limitativo di bilanciamento tra circostanze, tant'è che l'Italia già si era adeguata alla procedura di infrazione 2019/2033, con la quale la Commissione europea contestava il non corretto recepimento della direttiva relativa alle norme minime per la definizione dei reati e delle esenzioni nel settore degli attacchi contro il sistema di informazione. Il problema, quindi, non è circoscritto al sistema penale, bensì a quello culturale. L'ultimo punto critico relativo all'inasprimento sanzionatorio attiene alla materiale attuazione di quanto predisposto. Gli attacchi *hacker*, signor Presidente, avvengono per la maggior parte da Paesi terzi rispetto all'Unione europea. Questo lo abbiamo detto anche più volte in Commissione. Basti pensare che quelli attuati dai filorussi sono aumentati del 30 per cento nel corso dell'ultimo anno. Come pensa questo Governo di riuscire a colpire tali autori, considerate da un lato le sofisticatissime tecniche delle quali si avvalgono e dall'altro il luogo di commissione del reato, ovvero Paesi sui quali l'Italia non esercita alcuna giurisdizione? Un ulteriore tema è quello dell'invarianza finanziaria e qui torniamo al metodo. Non si vuole investire sulla cultura volta al contrasto della cybersicurezza: può pensare di combattere menti eccelse quali quelle degli *hacker* con investimenti pari a zero? Come si può pensare che il responsabile per la cybersicurezza possa intervenire se non si investe nella sua formazione? può pensare che un'agenzia governativa, auspicabilmente spogliata da magliette celebrative di congressi politici, possa adeguatamente fronteggiare tali minacce solo con i proventi derivanti dalle sanzioni? Ah, dimenticavo: anche con i tanto vituperati - dalla maggioranza, chiaramente - fondi del PNRR, reperiti grazie al Governo Conte. Servono investimenti. Il problema dell'invarianza finanziaria del provvedimento si riscontra anche in relazione a quanto accaduto in corso di esame alla Camera: se da un lato, infatti, si è introdotto un meccanismo volto a consentire le ispezioni ministeriali negli uffici giudiziari al fine di verificare la regolarità degli accessi alle banche dati, con evidenti rischi in materia di segretezza delle indagini, dall'altro proprio in ragione dell'obbligo di invarianza finanziaria è stato espunto dal testo il tracciamento dell'utilizzo delle banche dati pubbliche, un cortocircuito difficilmente spiegabile, visto che il provvedimento in questione era sorto proprio al fine di evitare che casi come quello ultimamente occorso si possano ripetere. Il Governo continua pervicacemente a perseguire, sin dal lontano decreto-legge di istituzione del delitto di *rave party*, logiche solo ed esclusivamente punitive. Serve invece investire sulla creazione di una cultura della cybersicurezza al fine di implementare una generalizzata consapevolezza dei rischi ai quali cittadini e imprese sono esposti. Quindi, non facciamo i soliti provvedimenti di facciata e - diciamola tutta - solo politicamente utili, ma entriamo nel cuore del problema ed affrontiamolo con la dovuta attenzione. Presidente, sicuramente il mio appello resterà, come al solito, disatteso e qui, da buona napoletana, mi vien da dire: «*A lava' a capa 'o ciuccio se perd' l'acqua e 'o sapone*». Grande saggezza napoletana. Invito la maggioranza e coloro i quali non avessero capito il significato del famosissimo e usatissimo proverbio napoletano, ad andarlo a vedere. *(Applausi)*.

Secondo i dati del rapporto annuale dell'Associazione italiana per la sicurezza informatica, il settore più attaccato in Italia è quello governativo-militare, con il 19 per cento degli attacchi, un incremento del 50 per cento rispetto al 2022, seguito poi dal settore industriale, in particolare quello manifatturiero, quindi di particolare interesse per il nostro Paese, con il 13 per cento, ed un incremento del 17 per cento rispetto all'anno precedente. Si capisce quindi immediatamente come i cyberattacchi vadano a colpire dei settori strategici del nostro Paese e non solo. In un momento in cui lo scenario geopolitico rischia di creare delle fragilità e delle vulnerabilità importanti, evidentemente non possiamo non rispondere con estrema fermezza ed è in questa direzione che vanno sia questo disegno di legge, sia le attività del Governo che finalmente affrontano la problematica offrendo soluzioni politiche e legislative, andando a creare quegli strumenti e anche, oserei dire, quella cultura per il rafforzamento delle difese *cyber.* E il riferimento fortemente voluto dalla Presidenza italiana all'importanza della cybersicurezza, fatto proprio nell'ultimo G7, ne è un'ulteriore dimostrazione. I dettagli del disegno di legge sono già stati adeguatamente illustrati e non vorrei in questo caso ripetermi, ma ci tengo a sottolineare alcuni aspetti che, secondo me, sono particolarmente significativi. Il Governo italiano ha promosso per la prima volta all'interno del G7 un gruppo di lavoro sulla sicurezza cibernetica, presieduto dal prefetto Frattasi, che è direttore dell'Agenzia italiana per la cybersicurezza nazionale, riunendo così tutti i responsabili delle agenzie e dei centri di responsabilità della cybersicurezza dei sette Paesi: il Canada, la Francia, la Germania, il Giappone, l'Italia, il Regno Unito e, non da ultimi, gli Stati Uniti. Importante iniziativa a trazione proprio italiana, che evidenzia la necessità di una maggiore cooperazione, ma anche di un maggiore coordinamento tra gli alleati e questo specialmente in un momento delicato a livello internazionale come quello che stiamo attraversando. Inoltre, il tema della cybersicurezza ha un valore anche, a nostro parere, strategico: la protezione la protezione da attacchi cibernetici dei nostri *asset* nazionali. Proprio le ultime crisi internazionali hanno dimostrato la pericolosità della cosiddetta guerra ibrida, poiché accanto alle minacce cosiddette tradizionali e provenienti dai domini classici come quello terrestre, quello aereo e quello navale, si sono aggiunte altre tipologie di azioni ostili ibride, provenienti dal cyberspazio, dallo spazio o con azioni, come sappiamo, di interferenza. Per questo, considerando l'ampliamento del concetto di minaccia alla sicurezza nazionale, è necessario rafforzare le difese sia tradizionali che ibride, e armonizzare il sistema Paese proiettato verso interno e l'esterno, proprio per innovarlo, migliorarlo, rafforzarlo e far crescere il peso specifico del nostro Paese nei consessi internazionali. E proprio sulle minacce ibride e sulle ingerenze esterne va ad includere la mia proposta, peraltro condivisa anche da alcuni colleghi sia di maggioranza che di opposizione, per discutere ed analizzare sul piano politico, attraverso gli strumenti che i Regolamenti parlamentari ci consentono, come rafforzare queste sfide. Dobbiamo dare per assodato che certe attività cibernetiche di potenze ostili siano evidentemente sinergiche alla destabilizzazione anche di nostre infrastrutture sensibili e strategiche; con uno scenario geopolitico in continuo mutamento, questo è un tema che non possiamo non affrontare. Proprio come questo Governo ha voluto tracciare la rotta, è necessaria una maggiore cooperazione non solo tra gli Stati europei, ma dell'intero Occidente. Rafforziamo la cooperazione con i nostri storici alleati, gli Stati Uniti, Uniti, ma anche con il Regno Unito, con Paesi amici come Australia, India, Taiwan, che - lo ricordo - anche per esperienze dirette sanno bene come affrontare gli attacchi cibernetici provenienti, ad esempio, nel caso di Taiwan, dalla Cina o dalla Corea. Rafforziamo inoltre quella cooperazione con le organizzazioni internazionali, come ad esempio la NATO, su questa tematica. Ritengo infine che solo con l'unità dell'Occidente potremo fronteggiare queste minacce ibride e difendere le nostre infrastrutture sensibili e strategiche, ma - lo voglio sottolineare - anche le nostre imprese ed aziende, poiché quando si parla di cybersicurezza non si parla solo di informatica in senso stretto, ma di vera e propria sicurezza nazionale. Signora Presidente, stiamo discutendo di un provvedimento importante che sta esattamente nell'attualità che stiamo vivendo e attraversando per tutto quello che attiene ormai all'evoluzione dell'informatica: oggi stiamo discutendo molto anche di intelligenza artificiale e, tra l'altro, la cybersicurezza

ha riconosciuto l'importanza e l'urgenza (d'altra parte anche nei Governi precedenti vi sono stati numerosi interventi in tal senso), ma ha voluto dare un poderoso contributo sia alla Camera che qui al Senato con degli emendamenti. Dal sottosegretario Mantovano, che si era reso protagonista di questa iniziativa legislativa, erano state date assicurazioni e rassicurazioni sul fatto che il contributo dell'opposizione sarebbe stato tenuto molto presente. Questo si è realizzato solo in piccola parte. Devo dare atto alla Sottosegretaria oggi presente in Aula, che sicuramente non si è risparmiata; è stata molto attenta ed ha ascoltato le nostre istanze. A un certo punto il sottosegretario Mantovano si è anche fisicamente eclissato e quindi permangono una serie di problemi e di perplessità, perché qui l'approccio ormai è sempre il solito: di fronte a una questione molto rilevante, sociale o tecnologica come in questo caso, di sicurezza nazionale e internazionale che sia, si fanno una serie di norme perlopiù punitive o di organizzazione senza senza affrontare il nodo del problema. Da un lato, vi è infatti la questione delle risorse, perché quando parliamo di modernizzazione e di essere all'altezza di un'evoluzione tecnologica che ha una ha una velocità più che supersonica (una volta abbiamo detto che va alla velocità della luce, ma ormai siamo molto oltre anche la velocità della luce), c'è una questione enorme di investimenti e di organizzazione. Vorrei intervenire sui due argomenti: uno è quello delle risorse invariate e l'altro è quello delle cosiddette ispezioni direttamente dipendenti dal Ministero della giustizia. Non si può dire che si affronta un problema di questo tipo a risorse invariate. Non lo si può dire, come

che il Governo, in particolare con il ministro Fitto, si sta impegnando per spendere efficacemente i fondi previsti a tal fine. Ma cosa vuol dire che si sta impegnando? Non si può

l'abuso d'ufficio; poi però, quando si tratta di dare loro le risorse per affrontare i temi, purtroppo non ce ne sono. Addirittura abbiamo appreso che, ai Comuni che sono stati bravi a fare i progetti per il PNRR, si tolgono le altre risorse che dovrebbero arrivare. È veramente un grandissimo paradosso. Vorrei ricordare che negli altri Paesi, per esempio negli Stati Uniti, su 65 miliardi di investimenti nel digitale, sono stati investiti 11 miliardi solo sulla cybersicurezza.

Per l'ennesima volta taglieremo sui servizi essenziali, perché c'è un problema di sicurezza. Qui c'è davvero un *deficit* di impostazione, e vorrei dire anche di serietà, nell'affrontare i temi della sicurezza. L'Italia è sicuramente indietro, come lo sono anche altri Paesi (ma l'Italia lo è sicuramente di più). Non possiamo non metterci Come dicevo, sono stati dati una serie di compiti agli enti locali e finanche alle aziende, quelle aziende che devono attuare una serie di disposizioni e alle quali avete detto: potete accedere ai bandi

che deve essere recepita e che è molto importante. Invece di aspettare per recepire questa direttiva, ci è stato detto che si farà più avanti, ad ottobre. A me spiace constatare, ancora una volta, che la tecnica dello sbandieramento delle norme, quando c'è una questione o un problema che ci preoccupa assolutamente tutti, è una tecnica che vale per tutto. E veniamo alla questione delle ispezioni, che è evidente, anche sull'onda di fatti di cronaca che hanno assolutamente preoccupato tutti. Immagino quali saranno gli interventi: è stata messa in pericolo la sicurezza delle persone con ingressi indebiti. Ma qui c'è un punto fondamentale. Voi date un potere ispettivo a un organo che dipende direttamente dal Ministero della giustizia, cioè è alle dipendenze di un organo politico, il quale potrà, esercitando un potere delicatissimo, entrare direttamente nella segretezza delle indagini in corso. Sarebbe fin troppo facile - un gol a porta aperta - ricordare che non abbiamo avuto delle prove così egregie di rispetto della segretezza di indagini, perché è recente e ancora non risolta, nonostante

politico. Tra l'altro, ricordando un argomento che ha sollevato in Commissione il senatore Scarpinato, con le modifiche che sono state fatte dalla legge Cartabia, oggi prima di iscrivere - giustamente, è una norma

siccome, per poter fare questo tipo di ispezione, devi innanzitutto vedere se sono iscritte notizie di reato e perché, noi faremmo sì che un organo politico entri direttamente, con tutti i piedi, nelle indagini in corso. Cosa ci voleva a prevedere altri tipi di controllo

poteri e tutto si tiene con la discussione che stiamo facendo in questi giorni anche sul premierato. Voi volete riscrivere non solo la Costituzione, ma anni e anni

cambiato il modo di attaccare gli Stati nazionali e di creare vere e proprie azioni di disturbo e di danneggiamento, capaci di mettere a rischio la sicurezza di una Nazione. Oggi più che mai occorre essere pronti, anche alla luce dei delicatissimi equilibri mondiali, a resistere ai cyberattacchi e a trovare adeguate contromisure per tutta l'area della sicurezza dei cittadini. Occorre quindi adeguare il portato normativo con un'esigenza di sicurezza che vada oltre il 2.0 e che ha rilevante impatto anche per l'economia della nostra Nazione. Per questo motivo è importante, signor Presidente, l'approvazione del provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea, per consentire all'Italia di dotarsi al più presto di strumenti che, per quanto le opposizioni possano dirsi non pienamente soddisfatte, sono certamente più adeguati di quelli attuali. Peraltro, la sicurezza cibernetica - e fughiamo il campo da ogni dubbio - è uno dei principali interventi previsti dal PNRR nell'ambito della trasformazione digitale, della pubblica amministrazione e della digitalizzazione del Paese. Quindi, si va nella direzione di prevedere una *governance* centralizzata degli aspetti di sicurezza e nuove disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati informatici. che compongono il disegno di legge, rispetto ai diciotto della versione originaria, grazie - va detto - all'approvazione delle proposte arrivate anche dall'opposizione nel corso dell'esame delle norme nelle Commissioni affari costituzionali e giustizia sia alla Camera sia al Senato. Per comprendere l'importanza dell'approvazione unanime di questo provvedimento, riporto i dati più recenti forniti dallo stesso sottosegretario Alfredo Mantovano in audizione: nel 2023, l'Agenzia per la cybersicurezza istituita dal Governo Draghi ha trattato 1.411 eventi (circa 117 al mese), con un notevole incremento rispetto ai dati del 2022. Per essere chiari, colleghi, per "evento" in questo caso si intende un avvenimento che ha un impatto su almeno un soggetto nazionale e che comporta un *alert* e un successivo intervento di rimedio nei confronti dei soggetti colpiti. L'altro lato sul quale occorre riflettere è quello fornito in audizione dal Direttore del servizio di Polizia postale e delle comunicazioni, che ci ha comunicato che l'Interpol stima in 10,5

con nuove disposizioni che riguardano la resilienza della pubblica amministrazione e del settore finanziario, i contratti pubblici di beni e servizi informatici impiegati a tutela degli interessi nazionali strategici, il contrasto ai reati informatici e la sicurezza delle banche dati degli uffici giudiziari. Tra i punti più qualificanti del disegno di legge c'è l'obbligo di segnalazione entro ventiquattr'ore all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di alcuni tipi di incidenti che hanno impatto sulle reti. A definire il perimetro di quest'obbligo, e quindi quali saranno gli enti pubblici e privati tenuti alla segnalazione, sarà la Presidenza del Consiglio, su proposta del Comitato interministeriale per la cybersicurezza. Altra novità introdotta dal disegno di legge è la disposizione che alle riunioni del Nucleo per la cybersicurezza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale potranno partecipare su specifiche questioni di particolare rilevanza i rappresentanti della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e della Banca d'Italia. Il disegno di legge prevede, tra le nuove disposizioni introdotte, che nelle pubbliche amministrazioni che ancora non l'abbiano fatto venga istituita una struttura *ad hoc* per la *cybersecurity* che si doti di un referente unico.

Anche questo ha a che fare con la cybersicurezza e con la rete di protezione che dev'essere costruita attorno alle banche dati, alle loro interrogazioni e all'uso che gli stessi dipendenti pubblici amministratori ne fanno. Nel caso emerso, sono venute fuori oltre 5.000 interrogazioni dei sistemi informatici in tre anni alle banche dati Serpico e Siva e la maggior parte delle interrogazioni è avvenuta a ridosso di elezioni politiche o ha anticipato indagini giudiziarie, fornendo *assist* ai giornali e ottenendo in cambio una sorta di sponda. fatti gravissimi, su cui sono in corso indagini e che debbono necessariamente fare riflettere, perché ci sono in ballo la sicurezza nazionale - è vero - ma anche la vita delle persone e il diritto alla riservatezza. Per questa ragione, tra i suoi articoli, il disegno di legge stabilisce anche le norme per l'accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni da parte degli addetti tecnici, prevedendo precisi sistemi di autenticazione. Secondo le nuove norme, i dipendenti che abbiano partecipato a specifici programmi di specializzazione non potranno assumere per almeno due anni incarichi presso soggetti privati con mansioni relative alla *cybersecurity*. Secondo le disposizioni del Capo II del disegno di legge viene introdotta e definita una serie di reati informatici grazie alla modifica di alcuni articoli correlati al codice penale, dall'accesso abusivo a un sistema informatico telematico alla detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico. introdotte aggravanti sulla truffa (aggravata, quindi), prevedendo la confisca obbligatoria di beni e strumenti informatici o telematici utilizzati in tutto o in parte per la commissione del reato, oltre che i profitti o il prodotto di questo genere di reati. Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge in questione prevede anche che venga punita la fattispecie del delitto di estorsione mediante reati informatici e l'innalzamento della pena per il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, che potrà costare da due a sei anni di reclusione. Il provvedimento prevede che i proventi delle sanzioni vengano indirizzati all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Tra le modifiche più recenti vi è la possibilità gli ispettori del Ministero della giustizia di fare controlli sull'accesso alle banche dati. Non possiamo più permettere il ripetersi di situazioni odiose, che minano la riservatezza della gente, di chi fa politica, di chi è un personaggio pubblico, per eventuali torbidi interessi. Non sarebbero azioni permesse in un Paese civile qual è il nostro e di certo non sono azioni che questo Governo potrebbe tollerare, poiché si è posto sempre in equilibrio e con garanzia per quanto concerne i diritti individuali. Le nuove disposizioni migliorano la resilienza delle infrastrutture critiche, promuovono l'adozione di tecnologie avanzate, come la crittografia, e rafforzano la cooperazione tra vari enti e servizi di sicurezza. I cittadini italiani devono essere tutelati. Il cybercrimine ha modalità operative infide e odiose e può causare pesantissime ripercussioni sulla vita delle persone. Non si può abbassare la guardia e per questo abbiamo innalzato un muro più robusto, creando un quadro normativo maggiormente aggiornato e adeguato alle nuove sfide del cyberspazio, costruendo un ambiente digitale più sicuro, protetto per le istituzioni, le imprese, i cittadini italiani. *(Applausi)*. A chi parla di scarsità, occorre ribadire che oggi il punto non è tanto aggiungere risorse ai 50 milioni di euro già stanziati per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, già previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, indirizzare, grazie a provvedimenti normativi come quello di cui oggi discutiamo, quelle risorse già esistenti in chiave preventiva. La prevenzione, quindi, costituisce un primo e importante *asset* in questa battaglia, per rafforzare la cybersicurezza e sensibilizzare enti e imprese affinché sappiano da dove possono venire le minacce, con l'obiettivo di fornire una guida concreta per la prevenzione, il rilevamento precoce, la risposta efficace e la ripresa rapida in caso di attacchi informatici. Questo testo, arricchito dagli emendamenti che sono stati approvati in Commissione e che verranno approvati tra breve, rafforza tanto la risposta penale alla minaccia alla sicurezza informatica, quanto la capacità di risposta della pubblica amministrazione. Concludo, Presidente e onorevoli colleghi, con una riflessione: per vincere la sfida della cybersicurezza e per contrastare la cybercriminalità occorrono norme adeguate, tecnicamente performanti ed efficaci, e soprattutto diffondere, ad ogni livello istituzionale,

Signor Presidente, intendo intervenire per porgere un ringraziamento da parte del Governo, in particolar modo da parte del sottosegretario Mantovano, ai Gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione, che, sia al Senato che alla Camera, hanno mostrato un atteggiamento di grande responsabilità rispetto a un provvedimento che tutti riteniamo urgente e affronta questioni allarmanti. Siamo tutti consapevoli

ringrazio davvero il Parlamento, perché non soltanto ha agevolato un *iter* spedito per l'approvazione di queste norme, ma ha anche contribuito realmente al miglioramento del testo, che addirittura oggi è superiore in termini di efficacia rispetto a quello proposto nella stesura iniziale. Ho ascoltato gli interventi, che sono stati, per certi aspetti, critici, perché hanno sollevato alcune questioni ovviamente non sono completamente risolte. Il provvedimento in esame non ha l'ambizione di avviare, sviluppare e concludere un percorso, perché la sfida cibernetica è molto complessa. Il provvedimento ha il merito di avviare e modernizzare dei sistemi di sicurezza che sono risalenti a vent'anni fa, e sappiamo fa, e sappiamo tutti che vent'anni per il *web* sono un'era geologica. Il Governo si ascrive questo merito e naturalmente lavorerà ancora tantissimo. Sul tema delle risorse siete intervenuti tutti. È stato un tema dibattuto.

come dotazioni dell'Agenzia disponibili attraverso i bandi PNRR, a cui potranno partecipare i soggetti ricompresi nel perimetro del disegno di legge. Lo sforzo del Governo sarà ulteriore perché è naturale che, dotando in futuro l'Agenzia di ulteriori risorse, altri strumenti e altri veicoli, queste norme saranno ancora più efficaci. C'è ancora tanto lavoro da fare e lo faremo. L'approccio è quello giusto. La collaborazione di tutti è auspicabile anche per il futuro. Ribadisco, quindi, i ringraziamenti da parte del Governo a tutto il Parlamento per l'ottimo lavoro svolto. Ho sentito anche qualche critica rispetto a norme accolte che forse non tutti sanno che sono state proposte dai Gruppi di opposizione. Mi riferisco in particolar modo a quella delle ispezioni che è stata proposta dal Gruppo di Azione e accolta dopo un ampio confronto tra Palazzo Chigi e il Ministero della giustizia. Vorrei rileggere il testo perché vedo molto allarme sul punto: «Nelle ispezioni è verificato altresì il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari». È una norma accolta da Gruppi di opposizione; è stata ampiamente affrontata e la riformulazione ha ridotto il rischio di indebito accesso alle banche dati da parte di persone non legittimate a farlo. È un'esigenza che evidentemente nasce a causa dei fatti di cronaca che tutti abbiamo ritenuto allarmanti e quindi, attraverso questo veicolo ripeto - dai Gruppi di opposizione, lo abbiamo affrontato nel miglior modo. Volevo fare quest'ultima precisazione. Vi ringrazio. Continuiamo a fare il buon lavoro che abbiamo iniziato a

c'è un'ispezione, si garantiscano il contraddittorio e il diritto di difesa. Quindi, chiediamo che chi viene coinvolto nell'ispezione sia messo nella condizione, come accade in ogni situazione,

un emendamento di sano buon senso, del tutto inoffensivo e in linea con i princìpi generali dell'ordinamento della Repubblica. Per questo mi stupisce il parere contrario. Chiedo un cambio di parere e, ovviamente, invito l'Aula e anche ai colleghi della maggioranza a votare per il nostro emendamento.

parere contrario su tutti gli emendamenti,

Grazie,

i quali sono abilitati, tramite credenziali, ad accedere alle banche dati e ai sistemi informatici e possono captare dati informatici coperti da segretezza per le finalità più varie: per fini di concorrenza industriale, finanziati da privati o da potenze straniere, per costruzioni di dossieraggio, per lucro. È quindi incredibile che il senatore Sallemi abbia citato il caso Striano, tuttavia il presente decreto-legge non preveda alcuna misura per prevenire e reprimere gli accessi indebiti da parte dei soggetti abilitati ad accedere ai sistemi informatici e alle banche dati. tanto più incredibile perché alla Camera dei deputati, siccome questo buco di sistema è stato individuato, le Commissioni competenti si erano messe d'accordo avevano previsto, appunto, che, per evitare questo problema, bisognasse elevare il sistema di accesso alle banche dati, prevedendo delle credenziali di accesso con dati biometrici, e soprattutto che dovesse essere previsto che tutti gli accessi effettuati alle banche dati dovessero essere sottoposti a un controllo sistematico successivo, mediante l'annotazione di chi aveva fatto l'accesso e delle motivazioni per cui era stato fatto l'accesso stesso. Ebbene, il 14 giugno la Camera dei deputati ha cassato questa parte della norma

difenderci dagli attacchi cibernetici, ma non abbiamo previsto assolutamente niente per difenderci contro i vari soggetti che, all'interno di tutte le banche dati nazionali e locali, in questo momento hanno la possibilità di accedere senza che che sia possibile, per via della mancanza di controlli successivi, verificare la regolarità dell'accesso. Quindi, abbiamo previsto un emendamento, che è lo stesso che era stato approvato dalla Commissione competente alla Camera, introduce la necessità che per accedere alle banche dati siano richieste credenziali di carattere biometrico e sia previsto un controllo successivo generalizzato a campione, a cadenza periodica, di tutti gli accessi effettuati. Abbiamo anche previsto che, per finanziare questa parte della legge, sia stanziata una somma di 10 milioni di euro da prelevare dal Fondo esigenze indifferibili. Mi sembra che non si possa - da una parte - citare il caso Striano e - dall'altra parte - poi proporre una legge che non ci difende assolutamente dalla ripetizione di casi simili. Speriamo, quindi, che questo emendamento venga approvato.

e della *privacy*, e quindi della riservatezza. Le tre cose vanno insieme ed evidentemente, se chi si occupa di *cybersecurity* non tiene conto anche degli aspetti legati alla *privacy* e alla transizione digitale, rischiamo che le pubbliche amministrazioni facciano una grande confusione.

Signora Presidente, signori del Governo, vorrei fare riferimento a due frasi per poi compendiare il senso dell'ordine del giorno presentato. La prima frase è stata pronunciata dal capo dei nostri servizi segreti, la dottoressa Elisabetta Belloni, il 28

se vogliamo mantenere le politiche liberaldemocratiche, dobbiamo mettere in atto politiche difensive sul versante della disinformazione. Un mese dopo, il nostro Capo di stato maggiore per la difesa e futuro presidente del Comitato militare per la NATO, l'ammiraglio Cavo Dragone, intervenendo nelle Commissioni congiunte di difesa e esteri di Camera e Senato,

è evidente che si contrappongono due visioni antitetiche della realtà e del mondo e noi non possiamo permetterci tentennamenti, perché ne vanno del nostro modello di vita e dei nostri valori democratici. Signora Presidente, signori del Governo e colleghi senatori, se il Capo dei servizi segreti e il Capo di stato maggiore della nostra Repubblica vengono in Parlamento e denunciano che c'è un problema legato alla disinformazione, alla sicurezza cognitiva e all'equilibrio delle fonti, questo Parlamento può chiudere gli occhi, far finta che non sia accaduto nulla e discutere di altro? A nostro giudizio, no. no. Se non bastassero poi questi allarmi che arrivano dai responsabili della nostra sicurezza, ci sono due ulteriori elementi che vanno nella direzione di rafforzare l'ordine del giorno che abbiamo presentato. Il primo: si è appena concluso il G7 e nel documento conclusivo è stato dato, giustamente, ampio spazio al tema dell'intelligenza artificiale generativa nel suo impatto sulla disinformazione, sulla misinformazione, sulla elaborazione di *fake news* in grado di impattare sulla formazione dell'opinione pubblica dei Paesi liberi. Ricordo che nei Paesi non liberi semplicemente queste cose non avvengono per note attività censorie da parte dei dittatori e delle dittature. Nell'ambito dei lavori preparatori del G7, il Governo italiano a Capri ha sottoscritto un protocollo d'intesa fra la Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America, sottoscritto dal ministro degli affari esteri Tajani e dal segretario di Stato Blinken, finalizzato a istituire attività contro la disinformazione per scopi militari e ostili nei confronti dell'alleanza occidentale. Da ultimo, non più tardi di ieri il nostro Presidente della Repubblica, in visita di Stato ufficiale in Moldova un tema e un posto non propriamente banale, anzi credo scelto appositamente per lanciare questo allarme - ha sollevato il tema della disinformazione, che mette a rischio la nostra sicurezza e i nostri *standard* democratici. Signora Presidente, siccome il contenuto di questo ordine del giorno è estremamente delicato, sul quale - a mio giudizio - le forze politiche non devono dividersi, ma devono trovare un punto di discussione e di convergenza, a fronte del parere contrario del relatore e del Governo ritiro il mio emendamento. Non voglio che ci sia un voto contrario dell'Assemblea

qualche perplessità rispetto al modo con il quale è stata liquidata, in sede di Commissione e oggi in sede di Aula, una tematica così importante come l'esigenza di costruire degli strumenti che tutelino la nostra libertà, la nostra libera informazione, i nostri standard democratici. Questo è comunque un elemento che deve essere preso in considerazione, perché altri Paesi che fanno parte del nostro sistema di difesa si sono dotati di questo tipo di strumenti. di strumenti. L'Italia, essendo uno dei Paesi dove è maggiormente presente un grado di disinformazione, in particolare condotto dagli strumenti e dalle piattaforme russe, come denotano i dati che si stanno diffondendo da parte di analisti e di centri di ricerca nel corso delle ultime settimane, deve prendere in considerazione con grande urgenza questi aspetti. Ritirando questo ordine del giorno, mi permetto però di sollecitare tutte le forze politiche e il Governo ad un approfondimento dovuto rispetto a una tematica che deve trovare un nostro necessario punto di approdo.

che si riferiscono - ne abbiamo parlato in Commissione con la sottosegretaria Siracusano - a una dotazione finanziaria che consenta a questo provvedimento di avere un senso.

dichiarazioni che cortesemente la Sottosegretaria ci ha reso in Commissione, che si riferiscono al PNRR e a successive fonti di finanziamento. Le prendiamo per buone come intenzioni; però dispiace vedere che un provvedimento così importante, rispetto al quale le opposizioni hanno avuto un atteggiamento estremamente collaborativo, come del resto la Sottosegretaria ha riconosciuto (anche di questo la ringrazio), sia privo dei fondi per le assunzioni e per la formazione, al fine di consentire a questo meccanismo di mettersi in moto. Noi, come opposizioni, non possiamo non notarlo; credo che il Governo lo comprenderà. Resta la disponibilità e resta la collaborazione, ma sul piano politico va sottolineato e detto in modo molto chiaro che questo provvedimento avrà una testa,

Signora Presidente, noi comprendiamo lo spirito dei pareri contrari, che sono volti a fare in modo che questa legge sia approvata tal quale, cioè, nella nella tradizione del nostro monocameralismo alternato, sia ratificata dal Senato come modificata dalla Camera. Però, diciamoci la verità, questi emendamenti gridano un po' vendetta. Quello che abbiamo appena votato parlava di un partenariato con l'università, per fare in modo che si creasse una cultura della *cybersecurity*, quindi interveniva a monte per fare in modo che le competenze tecniche necessarie a svolgere questi ruoli fossero create, appunto, a livello delle università. Invece, l'emendamento che andiamo a votare adesso si riferisce al sistema di valutazione delle prestazioni, che, come in ogni pubblica amministrazione, naturalmente dovrà essere implementato anche nell'Agenzia per la *cybersecurity*. Immagino che questo accadrà comunque, emendamento o non emendamento, perché un sistema di valutazione delle prestazioni deve stare necessariamente dentro ogni tipo di organizzazione, inclusa questa. Però, diciamoci la verità, se questo emendamento avesse avuto un parere favorevole e un voto favorevole da parte dell'Assemblea, avrebbe arricchito il testo e avrebbe avuto un suo senso.

Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

anche rispetto a intrusioni informatiche e non soltanto rispetto a quelle fisiche; quindi, se noi riteniamo che gli attacchi possano avvenire non soltanto nel mondo reale, ma anche in quello informatico, e stiamo applicando la normativa che applichiamo nel mondo reale, una volta ammesso che esiste un mondo digitale nel quale possono essere commessi reati,

che dovrà essere ovviamente proporzionato e necessario, così come avviene nel mondo fisico, deve essere considerato tale anche nel mondo digitale. Altrimenti si disarma, in un certo senso, la persona oggetto dell'attacco principale.

che è digitale, ma che esiste davvero, non è meno importante o meno seria. Allora, se la legge prevede che, in caso di attacchi fisici, la persona che subisce l'attacco possa, a certe condizioni, contrattaccare per legittimamente difendere il bene giuridico oggetto dell'attacco, dobbiamo necessariamente prevederlo anche nel mondo digitale. Per questo noi siamo molto preoccupati del parere contrario a questa proposta di modifica, che arriva anche dalla Camera dei deputati. Naturalmente voteremo a favore dell'emendamento, però sottolineiamo con forza la necessità che la norma vada in questa direzione.

a scenari che pongono il diritto penale, in particolare, dinanzi a sfide inedite, molto complicate e molto difficili.

si porrà ai giuristi e ai legislatori il tema di come combattere i reati che l'intelligenza artificiale può commettere. Pensiamo ai reati finanziari o ai reati connessi alle *fake news.* Sarà infatti molto complicato ipotizzare una responsabilità o una colpa per questi tipi di illeciti che verranno commessi, che saranno molto impattanti.

artificiale. Noi sappiamo che, per difendersi da questi attacchi, molto spesso - ne abbiamo parlato anche in Commissione con la Sottosegretaria - occorre, in qualche modo, attaccare a propria volta. Occorre cioè disabilitare i sistemi informatici che comportano gli attacchi informatici ai propri sistemi

sdoganare qualunque tipo di attacco preventivo che può diventare a sua volta un atto di pirateria. Bisogna trovare però il giusto bilanciamento tra la necessità di difendersi da questi attacchi e dalla pirateria informatica e il rischio di essere a propria volta sottoposti a procedimento penale perché si incorre negli stessi reati dai quali ci si vuole difendere.

Bazoli. L'accoglimento degli ordini del giorno evidenzia che il parere negativo sugli emendamenti non è una questione politica, ma tecnica. L'analogia fatta dal senatore Scalfarotto rispetto alla legittima difesa per un attacco fisico con armi è chiaramente suggestiva. Il rischio

abbiamo preso atto che questa maggioranza governativa, inspiegabilmente dal nostro punto di vista, sia alla Camera sia al Senato ha deciso di non introdurre alcun sistema per

nessun controllo, quindi, sugli accessi effettuati dai servizi segreti, nessun controllo sugli accessi effettuati dalle forze di polizia o dai funzionari dell'amministrazione statale, nessun controllo sui funzionari delle amministrazioni locali. Vi è una sola eccezione: questa maggioranza ha deciso che il pericolo viene da una sola categoria di funzionari dello Stato, cioè i magistrati, e ha previsto che solo per i magistrati debba essere svolto un controllo sugli accessi effettuati anche per le indagini in corso che sono coperte da segreto. Ha individuato questa categoria pericolosissima e ha introdotto una modifica all'articolo 7 della legge n. 1311 del 1962 che regola le ispezioni

può stabilire che vengano fatte delle indagini ispettive speciali anche su procedimenti in corso di svolgimento. Qui è stata introdotta la norma per cui l'ispettore ministeriale può effettuare controlli sugli accessi alle banche dati che sono state fatte dai magistrati. Come farà l'ispettore ministeriale a verificare se questi accessi alle banche dati sono regolari? Certamente non limitandosi a verificare il numero degli accessi effettuati, perché che siano dieci o cento poco cambia. Per verificare se questi accessi sono regolari, dovrà prima di tutto accertare su quali sono stati fatti tali accessi ed è evidente che, venendo a conoscenza dei nominativi delle persone sulle quali i magistrati che stanno indagando hanno fatto accessi, ci sarà la prima violazione del segreto investigativo. non basta, perché conoscere i nomi delle persone per le quali è stato fatto l'accesso non dice nulla; bisogna verificare se tale accesso è regolare e per farlo bisogna vedere se è pertinente alle indagini.

direttamente una persona perché c'è un sospetto; occorre che ci siano degli indizi tali da giustificare l'iscrizione. Ecco che, dunque, avremo squadernato tutte le indagini a un organo politico. Abbiamo pertanto previsto un emendamento emendamento soppressivo; tuttavia, se non accettate l'emendamento soppressivo, vogliamo almeno precisare che gli ispettori ministeriali non possono fare questi accessi quando c'è il segreto investigativo, cioè per le indagini in corso, e che possono essere fatti soltanto per le indagini non più coperte dal segreto investigativo? Se questo emendamento non verrà approvato, sarà chiara la volontà della maggioranza di introdurre un sistema che consenta all'organo politico di violare il segreto delle indagini e di sapere quali colletti bianchi sono indagati.

giorno G23.100, se accoglie la nostra sottoscrizione e per porre una riflessione, perché questa discussione è stata oggetto anche ieri dell'audizione del ministro Tajani in Commissione esteri ed è piuttosto curioso che il relatore chieda di espungere quel passaggio dell'ordine del giorno in cui si fa obbligo per il Ministero degli affari degli affari esteri e della cooperazione internazionale di rilasciare dichiarazioni formali attraverso i canali diplomatici in cui si afferma che il Governo prenderà di mira le organizzazioni criminali che lanciano attacchi *ransomware* a livello internazionale utilizzando alcuni strumenti di potere nazionale. Qui stiamo dicendo che il Ministero degli affari esteri non deve fare nulla. Vorrei che fosse chiaro: abbiamo previsto uno strumento legislativo per difendere il Paese da attacchi cibernetici che provengono per lo più dall'estero e il Governo ci ha detto che non dobbiamo occuparci della disinformazione - prendiamo atto - e che adesso, nel caso in cui registriamo che ci arriva un attacco di cybersicurezza dall'estero, il nostro Ministero degli affari esteri non deve fare nulla. Mi sembra che abbiamo una considerazione un po' particolare del modo con il quale dobbiamo difenderci.

abbiamo accolto la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno da parte del Governo e della maggioranza con la consapevolezza, naturalmente, che ciò che viene espunto avrebbe meritato ben altra attenzione, ma soprattutto considerando il fatto che il dispositivo è rimasto immutato.

Signor Presidente, onorevoli senatori, oggi ci troviamo ad affrontare un tema di cruciale importanza per la sicurezza nazionale e per la nostra società, la *cybersecurity*. Dispiace che questa discussione avvenga all'indomani del voto in Senato sul premierato e del voto di questa notte alla Camera, quindi inevitabilmente il Parlamento - non per questo momento ovviamente, ma in generale - è distratto rispetto a un tema che invece dovrebbe riguardarci molto da vicino. Gli attacchi informatici sono aumentati del 180 per cento rispetto a un anno fa.

Sono oltre 2.000 gli attacchi informatici al giorno, che mettono in una situazione di insicurezza quattro milioni di dati. Io penso che solo questi numeri dovrebbero essere motivo di riflessione. Molti di questi attacchi ovviamente vengono sventati, ma l'aumento è impressionante rispetto agli anni precedenti. E non si tratta di giovani *hacker* che operano per gioco o per provocazione, ma si tratta di professionisti e di esperti pagati talvolta da imprese straniere e altre volte da organizzazioni governative, quando non anche da Stati stranieri. L'Italia è tra i Paesi più esposti, con settori cruciali come il manifatturiero, i processi produttivi e i servizi socio-sanitari sotto costante attacco. Ecco perché riteniamo che la *cybersecurity* sia un tema di sicurezza nazionale ed europeo. Il Global information security workforce study ha stimato un *deficit* di competenze di 350.000 unità. Solo in Italia, secondo l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, servirebbero 100.000 esperti. Il Piano strategico nazionale, voluto dall'ex ministro Colao nel Governo Draghi e ora portato avanti dal Governo Meloni, prevede di spostare tutta la pubblica amministrazione sul *cloud*. Ma come possiamo trovare le persone che si occupino di *cybersecurity*? Come sa, Presidente, noi cerchiamo sempre, come Azione, di fare un'opposizione che non sia ideologica, ma che entri nel merito delle cose. Ci sono due temi in questo provvedimento che ci trovano favorevoli. Il primo è quello di riconoscere che il tema della *cybersecurity* è un tema di sicurezza nazionale ed europea. Il secondo è quello Il secondo è quello di chiedere che vengano estesi i soggetti (per esempio le società *in house*) che hanno l'obbligo di notificare tempestivamente gli incidenti che riguardano la *cybersecurity*. Cos'è che non ci convince di questo provvedimento? Sono due aspetti: il tema delle competenze, che è stato ricordato in tutti gli interventi delle opposizioni e che era presente in tutti gli emendamenti, e il tema delle risorse. risorse. Qualcuno pensa veramente, in quest'Aula, che basti individuare nella pubblica amministrazione un referente per la *cybersecurity* per aver risolto il problema della *cybersecurity*? Mi chiedo se veramente c'è qualcuno in quest'Aula che pensa che nominare un dipendente pubblico come responsabile della *cybersecurity* attenui il rischio di attacchi *cyber*. Mi chiedo dove pensiamo di poter andare, se vogliamo ridurre i rischi di esposizione agli attacchi *cyber* se non facciamo formazione. *(Applausi)*. Quando qualcuno mi dice Quando qualcuno mi dice che non ci sono le risorse, rispondo che non è vero e che le risorse a disposizione ci sono tutte. Il PNRR stanzia 623 milioni di euro per la *cybersecurity*. Quanti ne sono stati spesi fino ad oggi? 52 milioni, meno del 10 Non è vero che le risorse non ci sono; le risorse ci sono, è che non sappiamo utilizzarle. Come potremmo utilizzarle, per esempio, dal punto di vista della pubblica amministrazione? Noi abbiamo fatto una proposta molto semplice:

a disposizione una capacità di spesa di 300 milioni di euro l'anno, mentre noi spendiamo 5 milioni di euro l'anno per fare *reskilling*, cioè

che consenta ai giovani di entrare nella pubblica amministrazione per proteggere tutti i dati che mettiamo nel *cloud*? Sono dati estremamente sensibili per la nostra identità digitale. Eppure, rispetto a tutto questo, non abbiamo avuto alcuna possibilità di interloquire con il Governo, perché - come veniva detto prima - siccome il dispositivo è già passato alla Camera, noi sostanzialmente non possiamo che approvarlo così anche al Senato. Se noi non investiamo nella formazione e nel reclutamento di esperti e non utilizziamo le risorse messe a disposizione, non ci sarà mai quella prevenzione e quella efficacia che sono state richieste dai relatori e da esponenti della maggioranza. Solo così potremmo garantire la sicurezza dei nostri dati e delle nostre infrastrutture critiche. Per questo, come Azione, ci asterremo dal votare il provvedimento, perché di fronte a dei provvedimenti giusti, che erano anche in linea con ciò che veniva fatto precedentemente dal ministro Colao nel Governo Draghi, mancano le risorse e le competenze per rendere davvero efficaci le strumentazioni. Un'ultima annotazione di chiusura. Presidente, noi siamo in un contesto di conflitto, ci sono oltre 60 conflitti oggi nel mondo, ma attenzione che la *cybersecurity* interviene anche sul tema delle guerre cognitive, cioè su come si manipolano, attraverso la disinformazione e i dati, per preparare quei contesti che poi si affiancano a delle guerre cognitive, anche le guerre belliche. Non capire quanto sia strategico oggi il tema per la *cybersecurity* è una grave responsabilità. È il motivo per il quale, come Azione, ci asterremo da questo provvedimento. nell'ultimo decennio, con lo sviluppo tecnologico si è assistito ad un inarrestabile processo di

creando livelli di accessibilità delle informazioni e dei mercati prima impensabili, con una progressiva softwarizzazione della realtà. È come se il mondo avesse allacciato la sua spina alla Rete, collegandosi e abbattendo immediatamente le distanze. La rivoluzione digitale ha ridisegnato, tra l'altro, la logica e la struttura ingegneristica delle infrastrutture critiche degli Stati, divenute oggi totalmente dipendenti dalle soluzioni tecniche e digitali. Dai sistemi di gestione dell'energia e dell'acqua ai mercati finanziari e digitalizzati, dalla borsa telematica alla stessa pubblica amministrazione, agli ospedali, alle industrie strategiche nazionali: tutto oggi è basato sulla gestione e sulla condivisione dei dati, tanto che si parla di *digital continuum*, proprio come riferimento al fatto che, a prescindere dall'ambito di applicazione, la matrice di funzionamento è sempre basata sulla digitalizzazione e sulla condivisione e sullo scambio di dati. Ciò è stato agevolato, peraltro, dall'aumento esponenziale della capacità di calcolo dei computer, dalla crescita rapidissima di Internet; di contro, tuttavia, con lo sviluppo della Rete è anche cresciuta nel tempo l'azione malevola condotta attraverso di esse. Le autostrade digitali, che hanno messo in connessione gli utenti e anche costituito delle vie telematiche di accesso a sistemi di pregio, come siti governativi o *database*, contenenti informazioni di natura economico-militare, prima non erano accessibili, se non fisicamente. Ogni giorno la politica, l'economia e la finanza mondiali dipendono da Internet e dalle sue infrastrutture, per cui una manomissione o un attacco cibernetico potrebbero penalizzare settori nevralgici di un Paese, mettendo a rischio il funzionamento stesso dei servizi fondamentali e di interi apparati. Per dare una dimensione di concretezza a tale fenomeno, è utile evidenziare quanto riportato dal Rapporto Clusit 2024 sulla sicurezza ICT, che raccoglie i dati da fonti pubbliche, secondo le quali, negli ultimi cinque anni, la media mensile di attacchi gravi a livello globale è passata da 139 a 232. Se guardiamo all'Italia, la situazione è ancora più preoccupante, poiché, confrontando i dati del 2023 con quelli del 2019, emerge un aumento di attacchi *cyber* del 40 110 assalti informatici in un anno, di cui il 56 per cento di elevata gravità, come riportato dall'Associazione italiana per la sicurezza informatica. Si tratta principalmente del cosiddetto cybercrimine, anche se tra queste attività malevole se ne celano alcune che hanno una matrice non privata o isolata, bensì ben più radicate e riconducibili a organizzazioni statali, che utilizzano tali strategie per rallentare, colpire o disturbare il normale funzionamento di un Paese verso cui hanno un interesse contrapposto. Secondo quanto riportato nella relazione annuale 2023 sulla politica dell'informazione per la sicurezza, il progressivo ricorso ad armi digitali liberamente reperibili o distribuite sui mercati operando nel *dark web* da parte di gruppi criminali conferma verosimilmente la volontà dei Governi dai quali tali gruppi ricevono coordinamento tattico e strategico di conferire a quelle attività offensive la parvenza di comuni azioni criminali. La citata relazione evidenzia inoltre che nel 2023 è emersa una maggiore incisività delle azioni cibernetiche ostili di matrice spionistica poste in essere da gruppi statuali o sponsorizzati da Stati e si è ridotto il numero delle azioni di matrice non identificabile. La portata del fenomeno è spiegata dal fatto che un attacco cibernetico consente di ottenere effetti potenzialmente dirompenti a fronte di costi limitati e comunque di gran lunga inferiori rispetto a quelli necessari per organizzare, strutturare e mantenere aggiornato un sistema di difesa. Chi attacca riesce infatti a ottenere abbastanza facilmente risultati spesso anche eclatanti senza essere individuato, mentre chi subisce deve spesso lottare e prendere decisioni a più livelli, con incontri e riunioni di coordinamento, oltre che ovviamente con legislazioni nazionali spesso non adeguate e non ancora pronte a contrastare minacce di questo genere. A tal proposito, risulta fondamentale il lavoro svolto per il Paese con il disegno di legge fortemente voluto dal Governo e integrato in Parlamento in tema di disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici, che interviene con modifiche sostanziali e processuali, prevede, tra l'altro, l'introduzione del reato di truffa *online* con aggravanti per chi commette reati attraverso siti e piattaforme e fornisce un'adeguata risposta alle richieste tanto attese delle vittime, consentendoci di collocarci attivamente e con un aiuto concreto al fianco dei cittadini onesti e perbene. Sulla scia di tale importante provvedimento, è tuttavia fondamentale continuare ad agire bene e con urgenza per mettere in atto tutta una serie di iniziative sia organizzative sia strutturali, al fine di affrontare con la giusta determinazione e attenzione una questione tanto delicata soprattutto in una particolare fase della sicurezza internazionale come quella che stiamo vivendo, in cui ai conflitti internazionali si aggiungono le azioni spregiudicate condotte nel tempo della cosiddetta guerra ibrida. Non è un caso che la sicurezza cibernetica costituisca uno dei principali interventi previsti dal PNRR nell'ambito della trasformazione digitale della pubblica amministrazione e della digitalizzazione del Paese. È un esempio, a tal proposito, il rafforzamento voluto dal Governo delle funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ormai è l'attore principale della prevenzione e della gestione degli attacchi informatici. Certamente, tanto ancora si potrà e si dovrà fare, anche in termini economici, per supportare un'efficace strategia di sistema Paese in questo sfidante ambito, che - lo ricordo - è a tutti gli effetti un dominio operativo al pari di quelli terrestre, marittimo, aereo e spaziale. Mi riferisco, ad esempio, a iniziative quali *voucher* e crediti d'imposta per le aziende del comparto, crittografia nazionale per i servizi essenziali e decontribuzione specifica per le imprese del settore che assumono personale qualificato, oltre a specifici investimenti in tecnologie di nuova generazione dato valore aggiunto e in formazione del personale, elemento che rimane di fondamentale importanza anche in un contesto altamente digitalizzato come quello attuale. Tuttavia, sarebbe un grave errore ricondurre tutto solamente a previsioni di stanziamenti maggiori, in quanto molto si può ancora fare in termini sia organizzativi sia di *governance*. L'obiettivo è quello di unire le forze e le risorse, anche tecniche e umane, verso un sistema di cyberprotezione nazionale, basato su banche dati condivise e meccanismi di automatismo, di reattività, che permettano di accorciare il tempo che intercorre che intercorre tra attacco *hacker* e reazione, sì da preservare al meglio gli *asset*, le infrastrutture e le realtà economiche, politiche e sociali nazionali. Per essere competitivi nell'era moderna non è più sufficiente fare presto, ma occorre organizzarsi per anticipare gli eventi. Solo così si potrà mantenere l'iniziativa e si potrà avere un maggiore margine di successo. Ma anticipare su questi temi significa superare la pluralità di legittime posizioni di parte, nella ricerca di un obiettivo che non può che essere condiviso e perseguito da tutti con il massimo della convinzione e della forza.

che si intensificano particolarmente nei momenti elettorali attraverso alcuni siti permanenti, che lo fanno con maggior cautela, ma con evidenza, ma con una molteplicità di siti *web* che nascono e scompaiono velocemente. Una diffusa tempesta di disinformazione, di *fake news*, di falsità, volte tutte a screditare e destabilizzare, anche nel nostro Paese.

innanzitutto per esprimere il nostro rammarico rispetto alla decisione del Governo di respingere l'ordine del giorno del mio capogruppo, il senatore Borghi, su un'Agenzia che limiti la disinformazione. Infatti, se il Presidente della Repubblica decide di dire parole così nette, così chiare, abbandonando anche lo stile felpato che tradizionalmente caratterizza i messaggi del Quirinale, è perché la disinformazione non è più un sospetto: possiamo, a questo punto, considerarla un dato assolutamente accertato. C'è quindi innanzitutto un rammarico. Dall'altro lato, c'è un ulteriore elemento di rammarico, oltre a quello per il respingimento dell'ordine del giorno del collega Borghi, perché io credo che il Governo abbia perso una grande occasione di comprendere e poi spiegare al nostro Paese che il fenomeno della *cybersecurity* e il fenomeno della disinformazione sono in realtà due facce della stessa medaglia, sono praticamente la stessa cosa, la guerra cosiddetta ibrida, che si consuma, in particolare, tra la Russia e i suoi *partner*, da una parte, e il mondo libero, le democrazie liberali e il mondo occidentale, dall'altra. Si può tentare di attaccare in modo ibrido le democrazie liberali, ad esempio attaccando *server* con dati confidenziali, magari chiedendo un riscatto o, al limite, semplicemente rendendo pubblici i dati sensibili, come quelli sulla salute: abbiamo visto che è successo spesso e gli *hacker* che fanno questo tipo di operazioni spesso si trovano in altri Paesi. Oppure si può destabilizzare un Paese andando a influire sulla sua pubblica opinione. Noi sappiamo che purtroppo in Europa esistono forze politiche sensibili ai richiami del Cremlino, di Putin e dei suoi *partner* internazionali. Ricordiamo che in queste ore Vladimir Putin si trova a Pyongyang, con questo sancendo definitivamente il suo ingresso nell'esclusivo club degli Stati canaglia. Se vogliamo difenderci dalle minacce che arrivano dalla Rete e dal mondo digitale, noi non possiamo occuparci solo di una delle due questioni, ma dobbiamo occuparci di entrambe. Il fatto che questo disegno di legge non si occupi di questa parte io credo ne depotenzi grandemente la portata e il significato.

rendendosi conto poi di non avere le risorse. Oggi in quest'Aula venivano richiamati il nuovo Patto di stabilità e i 20-22 miliardi che bisognerà reperire per partire proprio con la scrittura della legge di bilancio che andremo a esaminare a fine anno. Purtroppo c'è da dire che questo disegno di legge, come tante altre misure, non ha fondi. Ho già detto nella fase di discussione, interloquendo con la sottosegretaria Siracusano, che comunque ringrazio moltissimo per il lavoro svolto, che è un punto di grande differenza nella visione del Governo e in quella di questa opposizione. Noi riteniamo questo disegno di legge poco più che un'elaborazione di buoni propositi, di desideri. Se si vuole combattere una cosa così complessa come la minaccia informatica,

di momento in momento. Non si può tentare di opporsi alla minaccia cibernetica con un approccio burocratico, con un manuale cartaceo di 500 pagine che ti dice cosa fare e in quale momento. Bisogna essere capaci di intervenire in modo efficace rincorrendo una tecnologia che quotidianamente si modifica e che, anzi, chi utilizza questa tecnologia in modo malevolo sa bene di dover rendere sempre più complessa. È una sorta di rincorsa; da un lato, vi è la minaccia che diventa sempre più difficile, insinuante e capace

di prevedere e vedere arrivare in anticipo le possibilità tecniche di far fronte a questa minaccia. Senza soldi tutto questo non è possibile. Diciamoci allora la verità: finché non vedremo delle risorse concrete e notevoli dedicate a questo intervento, penseremo che si tratta soltanto di un pannicello caldo. C'è poi un ulteriore elemento che è un po' il *fil rouge* del modo di operare del Governo ed è quello che quando c'è un problema, quando c'è qualcosa che allarma l'opinione pubblica, una bella norma penale non si nega a nessuno. Signor Presidente, le parlo da componente della Commissione giustizia, ormai sono quasi due anni che sforniamo senza sosta norme penali, nuove pene e manette, con il risultato, di cui abbiamo parlato anche ieri in quest'Aula, della situazione drammatica delle nostre carceri per il loro sovraffollamento. Abbiamo visto che ormai anche la giustizia minorile è stata equiparata sostanzialmente a quella degli adulti ed anche i ragazzini finiscono sempre di più nelle carceri.

delle norme che sono proprie del mondo reale al mondo digitale richiede che poi si pongano anche le garanzie che noi mettiamo nel mondo reale a tutela, per esempio, di chi si difende da un attacco anche nel mondo digitale.

è una disamina severa, che farebbe pensare a un voto contrario. Invece, devo dire che, come tutte le altre opposizioni, anche noi ci asterremo, perché capiamo

del fatto che tutte le opposizioni si sono comportate responsabilmente, come anche il Sottosegretario ha riconosciuto, sia in sede di Commissione che di Aula, è però giusto lasciare agli atti quelle che sono le carenze e i problemi che restano in piedi. Quindi, dando prova, ancora una volta, di grande responsabilità, il nostro sarà un voto di astensione, ma che non può non sottolineare un atteggiamento di seria critica al modo di lavorare del Governo, che abbiamo visto in questi due anni e che vediamo, di fatto, anche in questo provvedimento. *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, come Alleanza Verdi e Sinistra esprimiamo oggi una certa preoccupazione riguardo al provvedimento in discussione in Aula, già approvato alla Camera e volto a rafforzare la cybersicurezza nazionale. Sebbene, ovviamente, condividiamo le finalità del disegno di legge, notiamo, però, criticità nelle modalità con cui si intende raggiungere questi obiettivi e alcune carenze non colmate durante la discussione alla Camera. La sicurezza informatica è un tema imprescindibile, reso urgente dall'aumento di attacchi mirati a disabilitare sistemi informativi o a estrarre dati fraudolentemente. Siamo d'accordo, ovviamente, sulla necessità di di un intervento regolamentare e operativo per rafforzare le difese cibernetiche. Tuttavia, nel testo attuale notiamo diverse problematiche. La prima criticità, come hanno sottolineato un po' tutti i miei colleghi, è l'assenza di fondi. Non si può implementare un provvedimento di questa portata a costo zero. Inoltre, manca chiarezza sulla formazione *cyber* dei dipendenti pubblici, come faceva notare il collega Lombardo, e sarebbe necessaria l'assunzione di esperti specifici in materia di cybersicurezza. Il provvedimento si concentra principalmente sull'aumento delle sanzioni amministrative e penali che, sebbene possano avere un effetto deterrente, non sono sufficienti a prevenire atti illegali, soprattutto quelli compiuti all'estero. Le sanzioni arrivano spesso troppo tardi, quando il danno è già fatto. L'aumento delle responsabilità per le pubbliche amministrazioni e altri soggetti privati senza corrispondenti risorse economiche per formazione e acquisizione di competenze è un ulteriore problema. Signor Presidente, l'Italia è il fanalino di coda del G7 nel rapporto tra spese per cybersicurezza e PIL, nonostante l'impegno del Governo a investire l'1,2 per cento degli investimenti nazionali lordi in questo settore. Inoltre, nel provvedimento non sono adottati gli adeguati strumenti necessari per tutelare la particolare riservatezza dei dati custoditi presso gli uffici giudiziari. Questa è una lacuna che non si è voluta colmare, signor Presidente, e che lascia aperto uno spazio di pericolosa discrezionalità in mano a chi effettuerà i controlli. Ancora, sarebbe stato necessario un investimento economico nella formazione dei giovani e degli studenti per sensibilizzare sul tema della cybersicurezza e promuovere l'uso responsabile dei dispositivi digitali. Serve un intervento concertato con il Ministero dell'istruzione per integrare questi temi nei discorsi didattici. Siamo sorpresi che il Governo abbia affrontato il tema della cybersicurezza a costo zero. La cybersicurezza è una forma di difesa essenziale. Affrontare questa sfida senza un adeguato supporto finanziario rischia davvero di compromettere gravemente la nostra sicurezza informatica. Signor Presidente, questo provvedimento non ci piace e, alle nostre legittime preoccupazioni, questa maggioranza ha scelto di non rispondere. È per questo che noi di Alleanza Verdi e Sinistra voteremo no. Signor Presidente, sottosegretario Siracusano, onorevoli colleghe e colleghi, dopo un lungo e attento esame nell'altro ramo del Parlamento, arriva al vaglio di quest'Aula il disegno di legge di iniziativa governativa che ha per oggetto la cybersicurezza. Le questioni sul tavolo appaiono di strettissima attualità e di urgente approvazione. Il perimetro nazionale di *cybersecurity* deve infatti essere aggiornato e presidiato con la massima attenzione e con risorse adeguate e via via crescenti. Quanto sta accadendo sullo scenario strategico e geopolitico internazionale è sotto gli occhi di tutti e rende evidente che gli Stati nazionali devono ormai difendere i propri interessi e i propri confini non solo nello spazio fisico, ma anche in quello cibernetico. Guardiamo solo a quello che sta accadendo nella guerra russo-ucraina e nel conflitto di Gaza tra Israele ed Hamas. In questi teatri bellici le strategie di *cyberwarfare* e di *cyberwar* da parte di tutti i contendenti sono ormai sofisticatissime e si manifestano attraverso un'ampia gamma di azioni, dallo *hacking* per l'acquisizione di dati sensibili, fino al sabotaggio di sistemi vitali, passando per le campagne di disinformazione mirate ad influenzare l'opinione pubblica. La *cyberwarfare* si manifesta in modo eclatante nei tradizionali conflitti militari (abbiamo citato Gaza e l'Ucraina), ma purtroppo ormai viene attuata anche in tempo di pace apparente in forma anonima e clandestina, nell'ambito dello scontro epocale, sempre più aspro e pericoloso, che è in atto tra democrazie liberali occidentali e dittature o autocrazie orientali, con la finalità di indebolire gli apparati statali e alimentare scontento popolare e tensioni sociali. Anche il nostro Paese e le sue aziende strategiche, che non sono estranei al contesto internazionale, sono purtroppo costantemente nel mirino di *hacker* sempre più abili e sofisticati. Negli ultimi anni, proprio in coincidenza con il conflitto ucraino e quello a Gaza, gli attacchi si sono moltiplicati e sono diventati sempre più insidiosi, prendendo di mira anche le nostre infrastrutture energetiche, i Ministeri, gli ospedali e gli istituti finanziari. La difesa del dominio cibernetico richiede però un approccio multidimensionale, che va oltre la semplice protezione tecnica delle infrastrutture. Essa comprende la resilienza dei sistemi, la formazione di una cultura della sicurezza per gli utenti, la cooperazione internazionale per lo scambio di informazioni e strategie, nonché lo sviluppo di capacità di deterrenza credibili. A queste finalità tende appunto il testo di legge odierno, che aggiorna la legislazione interna per renderla il più adeguata possibile ai continui vorticosi sviluppi di una tecnologia in costante divenire. Il tema principale è dunque quello del rafforzamento della cybersicurezza nazionale. Ad esso sono collegati quello della resilienza delle pubbliche amministrazioni, del settore finanziario, del personale, del funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, dei contratti pubblici di beni e servizi informatici impiegati a tutela degli interessi nazionali strategici. Sono interventi assolutamente necessari, che dovranno essere attuati con la massima tempestività ed accuratezza dalle amministrazioni interessate, con la consapevolezza di un successivo incessante aggiornamento. Presidente, l'attualità non ci parla soltanto di attentati alle banche dati del nostro Paese ad opera di *hacker* internazionali al soldo di potenze straniere, per destabilizzare il quadro politico e a scopo di estorsione economica. Le cronache più recenti hanno, invece, portato all'attenzione dell'opinione pubblica e di questo Parlamento anche accessi abusivi alle banche dati ai fini di dossieraggio politico e di commercio di dati sensibili: un fenomeno gravissimo. di operazioni sospette (SOS) messo in evidenza dalla procura della Repubblica di Perugia dopo la denuncia del ministro Crosetto, che aveva visto pubblicati sulla stampa dei dati sensibili assolutamente riservati. In questo quadro è emerso, come ricorderà, signora Presidente, un numero spropositato di accessi abusivi da parte di un finanziarie infedele distaccato presso la Procura nazionale antimafia, che hanno riguardato tantissimi politici, sportivi, personaggi dello spettacolo (tra gli altri anche la collega Stefani, molto stimata e che credo interverrà più avanti sullo stesso argomento). Sono stati ascoltati di fronte alla Commissione parlamentare antimafia, il procuratore della Repubblica di Perugia, dottor Cantone, e il procuratore nazionale antimafia, dottor Melillo, che hanno evidenziato gravissime criticità nella gestione e tutela delle banche dati. Dalle loro audizioni è emerso un quadro sconfortante: le nostre banche dati possono definirsi in buona sostanza un colabrodo. Tuttavia il caso specifico ha fatto emergere anche gravi carenze normative: l'attuale disciplina dei reati informatici appare inadeguata alle criticità emerse e prevede pene in effetti troppo blande. Noi di Forza Italia condividiamo, quindi, appieno la revisione del quadro normativo e anche l'inasprimento delle pene previste in questo testo di legge. Credo che sia noto a tutti in quest'Aula che in generale chi parla e l'intero Gruppo di Forza Italia rimane perplesso, se non critico, rispetto al fenomeno del panpenalismo, peraltro assai in voga negli ultimi anni, che comporta un significativo aumento di nuove fattispecie penali e delle pene. Almeno in questo caso, però, non possiamo che condividere la proposta del Governo di inasprire le sanzioni e di delineare e differenziare meglio le condotte penalmente rilevanti, perché si tratta di reprimere comportamenti la cui pericolosità sociale si sta dilatando a dismisura con il passare del tempo per il frenetico sviluppo delle nuove tecnologie. In questo, mi distinguo nella valutazione dal collega Scalfarotto che, sul tema del contrasto al panpenalismo, mi trova spesso in posizioni similari. Le novelle riguardano pertanto diversi articoli del codice penale e del codice di procedura penale che riscrivono l'intera disciplina della materia. È stata introdotta, tra l'altro, la previsione secondo cui l'ispettorato generale presso il Ministero della giustizia, nel corso dell'ispezione ordinaria, dovrà anche verificare il rispetto delle prescrizioni sull'accesso e l'utilizzo delle banche dati dei tribunali. Mi pare una norma del tutto ragionevole, la cui approvazione alla Camera è stata accompagnata da qualche polemica - ho sentito anche poc'anzi delle critiche che però non condivido da parte del senatore Scalfarotto - una norma di buonsenso e ragionevole. Il giudizio da parte del nostro Gruppo su questo disegno di legge, dunque, è assolutamente positivo e di conseguenza Forza Italia lo voterà con convinzione. In conclusione, mi permetta un'ultima considerazione, signor Presidente. operazione sospetta (SOS), cui abbiamo fatto cenno poc'anzi nell'intervento, pare sparito dall'agenda politica. Il caso ha riempito per settimane le pagine dei giornali; taluno è giunto a definirlo lo scandalo più grave negli ultimi trent'anni e ce ne siamo occupati anche in Commissione antimafia. Nel frattempo, il finanziere coinvolto ha rilasciato interviste televisive ai quotidiani, ma poi stranamente il caso è uscito dai *radar* e da qualche tempo di esso non si parla più neppure in Commissione antimafia.

il MoVimento 5 Stelle si asterrà dal voto perché questo disegno di legge gravemente inadeguato ad assolvere l'importante e urgente finalità di dotare l'Italia di una vera protezione cibernetica. Ci troviamo dinanzi a un disegno di legge che nasce con gravi carenze strutturali e che in larga misura è destinato a restare inefficace, perché si limita ad affrontare problemi sostanziali con soluzioni meramente formalistiche. Quanto alle carenze strutturali, mi limito a segnalare una tra le più evidenti e gravi: tutto il disegno di legge è concentrato esclusivamente sul potenziamento dei sistemi di difesa contro gli attacchi *cyber* esterni, ma non prevede nulla per prevenire gli attacchi interni, cioè le intrusioni occulte e illegali nei sistemi informatici e nelle banche dati da parte di operatori infedeli per acquisire informazioni coperte da segreto per finalità di varia tipologia, ad esempio acquisizione di informazioni e di segreti industriali per finalità di concorrenza sleale da parte di privati o da parte di potenze straniere; acquisizione di informazioni ai fini di dossieraggio o di lucro; intrusioni realizzate mediante la corruzione o la complicità di soggetti in possesso delle credenziali ufficiali di accesso ai sistemi informatici. Si tratta di una falla inammissibile che priva il sistema di ogni difesa adeguata contro forme callide e insidiose di captazione illegale dei dati. E appare per me incomprensibile l'intervento del senatore Zanettin, che ha impiegato vari minuti a ricordare lo scandalo Striano e poi approva un disegno di legge che non prevede alcuna misura di prevenzione e di repressione. *(Applausi)*. Ma di cosa stiamo parlando? Quanto alla inadeguatezza delle misure previste contro gli attacchi esterni, questo disegno di legge è destinato in buona misura a restare una legge manifesto, perché - da una parte - prevede nei primi quindici articoli una serie di oneri, di obblighi, di adempimenti a carico di amministrazioni centrali e locali e - dall'altra parte - con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 24 priva tutti i soggetti che sono stati onerati e obbligati delle risorse essenziali (personale qualificato, attrezzature, fondi) per assolvere a questi obblighi.

nell'istituire presso l'amministrazione centrale e locale la nuova figura del referente per la cybersicurezza, al quale viene assegnato un compito strategico, si ribadisce che l'incarico deve essere conferito nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Come si può ritenere che il responsabile per la cybersicurezza possa fronteggiare la sfida lanciata da *hacker* altamente specializzati se non si investe nella formazione; se non vengono neppure indicati i criteri di certificazione di tali soggetti; se non sono esplicitati i requisiti di professionalità; se non è prevista una procedura periodica di verifica delle loro attitudini e di capacità? Questa è una scatola vuota. L'articolo 10, che istituisce il Centro nazionale di crittografia, al quale viene assegnata la *mission* essenziale della promozione della crittografia per il rafforzamento dell'autonomia industriale e tecnologica dell'Italia, ribadisce che comunque il Centro deve essere istituito a costo zero, cioè nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. Potremmo continuare a lungo con questi esempi, ma sono sufficienti a capire che ci troviamo dinanzi a una scatola vuota o semivuota. Se il I Capo del disegno di legge si palesa assolutamente inadeguato per il carattere meramente formalistico e nominalistico di molte delle soluzioni adottate, il II Capo, quello dedicato al potenziamento della risposta penale per prevenire e sanzionare la comunità informatica, si rivela, a un attento esame, altrettanto inefficace per una pluralità di ragioni. Il potenziamento della risposta penale, infatti, nel disegno di legge viene realizzato con l'aumento delle pene per i reati informatici, sia per il minimo che per il massimo; con l'estensione, per alcuni dei più gravi reati informatici, della disciplina delle intercettazioni per i fatti di criminalità organizzata; con l'istituzione di forme di coordinamento tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l'autorità giudiziaria. È È evidente che l'aumento delle pene è destinato a non avere alcuna efficacia deterrente nei confronti degli *hacker* stranieri che operano sotto anonimato per finalità politiche, agendo da Paesi sui quali l'Italia non esercita alcuna giurisdizione o o dai quali non può attendersi realisticamente alcuna collaborazione ai fini delle indagini. Si dirà che arrestano i criminali informatici italiani e quelli europei, ma non è si tratta di soggetti che, in larga misura, sono dotati di un'eccezionale professionalità e spesso appartengono a strutture complesse. Tali soggetti, per non rendersi tracciabili e per immunizzarsi dalle intercettazioni vocali e telematiche della magistratura, utilizzano piattaforme di comunicazione crittografata e criptotelefonini che consentono la comunicazione vocale di messaggistica in forma cifrata. Ebbene, nel corso di un'audizione del 20 giugno 2023 dinanzi alla Commissione giustizia del Senato, il generale Pasquale Angelosanto, comandante del Raggruppamento operativo speciale dei Carabinieri, ha illustrato in modo dettagliato queste modalità di comunicazione criptate, spiegando che la magistratura e la Forza di polizia italiana sono impotenti a intercettare i criptotelefonini. L'Italia, a differenza di altri Paesi europei, come ad esempio la Francia, non ha investito le risorse necessarie per stare al passo con l'evoluzione tecnologica. Lo stesso generale ha riferito che le Forze di polizia italiane per condurre alcune importanti indagini sono state costrette a chiedere la trascrizione delle intercettazioni di telefonate effettuate con i criptotelefonini alla polizia francese, che invece si è attrezzata da tempo. La necessità urgente di investire risorse per colmare questo gravissimo *deficit* operativo della magistratura e delle Forze di polizia italiane è stata da tempo rappresentata al Ministro della giustizia anche dal procuratore nazionale antimafia. Ma il ministro della giustizia Nordio e questa maggioranza sono rimasti completamente inerti su questo fronte cruciale, perché in questi lunghi mesi hanno profuso tutte le energie e le risorse per un impegno ritenuto di carattere capitale e prioritario, ossia l'impegno di limitare in ogni modo le intercettazioni della magistratura nei confronti dei colletti bianchi che ancora non si sono attrezzati con i criptotelefonini. Ecco i risultati di una legge sulla cybersicurezza che pretende di fronteggiare la criminalità informatica con il "bau bau" dell'innalzamento di pene che non potranno essere applicate e con le pistole caricate a salve di strumenti di intercettazione inefficaci per la loro sopravvenuta obsolescenza tecnologica. In sostanza, anche per la parte penale si risponde a pericoli gravi e attuali, invece che con soluzioni reali ed efficaci, che richiedono un investimento di risorse, con la facile scorciatoia di un'illusione repressiva affidata a grida manzoniane destinate a restare La stessa inefficacia caratterizza l'innalzamento delle pene previste per il reato di accesso abusivo ai sistemi informatici e telematici, previsto dall'articolo 615-*ter* del codice penale - per intenderci, il reato che è stato contestato a Striano destinato a prevenire e reprimere gli accessi abusivi ai contenuti dei sistemi informatici e delle banche dati da parte di operatori infedeli dotati di credenziali di accesso. Tutti i criminologi sanno che non è la gravità delle pene comminate a disincentivare la consumazione dei reati, ma è il concreto rischio di essere scoperti e quindi puniti. Attualmente il rischio di essere scoperti, per gli operatori interni al sistema che effettuano accessi abusivi, è minimo, perché non esiste un sistema generalizzato di controllo a posteriori degli accessi che sono stati effettuati, per verificare con cadenza regolare la conformità di questi accessi a ragioni di servizio. Per rendere efficace la repressione penale degli accessi abusivi alle banche dati, occorreva dunque prevedere l'annotazione degli accessi eseguiti in appositi registri, unitamente alle motivazioni che li hanno determinati e alla descrizione sintetica delle operazioni svolte, e procedere quindi a un controllo a posteriori degli accessi eseguiti con cadenza regolare. Ma questa maggioranza parlamentare ha eliminato la parte della legge che consentiva questi controlli successivi. Si perpetua così - mi avvio a concludere - e si legittima ancora una volta, per mancanza di volontà politica di investire le risorse necessarie, una falla di sistema che che riduce ai minimi termini il rischio di essere sorpresi e scoperti per gli operatori infedeli più accorti, che non si lasciano certamente intimidire da norme penali ridotte a tigre di carta. una falla di sistema che si lascia in vita per tutte le pubbliche amministrazioni, con un'unica significativa eccezione che riguarda i magistrati. È stata infatti introdotta, con efficacia immediata, una norma *ad hoc* che attribuisce al Ministro della giustizia il potere di disporre, quando lo ritenga opportuno, ispezioni straordinarie e mirate negli uffici giudiziari per verificare gli accessi alle banche dati effettuate dai magistrati, anche per le indagini che sono in corso di svolgimento. Tenuto conto che in questi casi la regolarità degli accessi non può essere riscontrata con il semplice dato numerico degli accessi eseguiti, ma solo mediante la cognizione dei nominativi dei soggetti per i quali siano state effettuate delle ricerche sulle banche dati, al fine di verificare la pertinenza o meno di questo accesso con le indagini, è chiaro che abbiamo creato uno strumento straordinario per aggirare il segreto investigativo. La bocciatura, oggi in Aula, dell'emendamento che prevedeva che questa ispezione non poteva essere effettuata quando le indagini sono in corso dimostra la volontà di mettere in mano a un organo politico uno strumento per scoprire il segreto delle indagini. Concludo, ricapitolando: pochi spiccioli per potenziare le difese contro gli attacchi *cyber* esterni; zero investimenti per consentire le intercettazioni dei criptotelefonini e delle piattaforme criptate; zero investimenti

Presidente, onorevoli colleghi, i dati che sono emersi e sono stati più volte ricordati dai colleghi nel corso degli interventi penso non abbiano bisogno di essere ripetuti. È chiaro ed evidente che negli ultimi anni, e anche proprio recentissimamente nell'ultimo anno,

piuttosto preoccupante e di certo non è un fenomeno recente o appena nato. È un fenomeno che si è sviluppato chiaramente negli ultimi anni, anche grazie al progresso delle tecnologie,

Il problema è che molti degli attacchi che sono stati posti in essere hanno avuto degli esiti e hanno raggiunto il loro obiettivo. Molti di questi attacchi sono stati rilevati e faccio riferimento in particolare dell'Associazione italiana per la sicurezza informatica. Qui si parla anche di attacchi che vengono considerati di gravità critica o elevata. Tra gli ulteriori dati preoccupanti che uno dei settori più attaccati dai cosiddetti *hacker* in Italia è stato proprio quello governativo-militare. Tra l'altro, negli ultimi tempi, non si può non correlare questo tipo di attacco con una situazione di conflitto oltreconfine. Ma noi sappiamo bene che ormai le guerre che stanno interessando il mondo stanno riverberando i propri effetti anche all'interno del nostro Paese, così come si è visto nell'ambito delle questioni di approvvigionamento energetico, nel momento in cui è scoppiata la guerra russo-ucraina. settore che preoccupa e ha preoccupato molti i cittadini, perché per un verso magari si può non avere un'immediata cognizione della pericolosità di un attacco *cyber* sugli apparati militari o governativi; magari i cittadini non lo percepiscono subito, ma percepiscono molto di più quello che è un altro settore che è stato particolarmente oggetto di attacchi informatici, che purtroppo è il settore della sanità, tra l'altro con attacchi e minacce

Non si può non approvare l'intervento da parte del Governo, che veramente ringraziamo per questo disegno di legge molto importante e coraggioso, che è intervenuto proprio per dare una risposta massiva e organizzata nei confronti di un fenomeno preoccupante e pericoloso che difficilmente potrà essere subito arginato solo con un provvedimento, perché avrà bisogno di una serie di barriere e strumenti che dovranno essere messi in pista a breve nel futuro. Dovremo continuamente correre dietro a quella che è una tecnologia che spesso è in mano a bande criminali, purtroppo - e sottolineiamo sempre il nostro purtroppo - sono più veloci anche della politica, dei processi decisionali e anche di quelli che possono essere gli strumenti a disposizione di una pubblica amministrazione, la quale ovviamente lavora nell'ambito della legalità e non certo in quello dell'illegalità. Abbiamo avuto modo anche di approfondire questo tema sotto altri versanti in Commissione giustizia, in sede di indagine conoscitiva proprio sul mondo delle intercettazioni, e di capire come i sistemi in mano alla malavita sono spesso molto progrediti; lavorano anche su piattaforme

e di valorizzazione dell'Agenzia sulla cybersicurezza, che quindi dovrà essere il contenitore all'interno del quale fare collegamenti tali da permettere che, per

Chiaramente sono previsti un aumento e un innalzamento delle pene con riferimento anche all'attività che viene svolta da un incaricato di pubblico servizio o da un pubblico ufficiale, che, per applicarla anche al caso dell'accesso abusivo ai sistemi informatici,

sono informazioni preziosissime che possono essere utilizzate variamente, dal mero dileggio, comunque fastidioso, a ben più gravi prospettive, dal ricatto all'utilizzo su piattaforme diverse (parliamo anche di minori, per non dire altro). Importantissime poi sono le aggravanti previste nel caso in cui gli accessi abusivi vengano fatti su sistemi informatici di interesse militare inerenti alla sicurezza e soprattutto - come si diceva prima - alla sanità.

pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio, che abusar di una sua posizione, prevedendo un accesso, ad esempio con un'installazione abusiva di apparecchiature su sistemi informatici o telematici, o fa intercettazioni illecite su conversazioni telefoniche.

ci troviamo di fronte - come vediamo adesso - problemi veramente importanti del nostro Paese, a cui occorre dare una risposta. La Lega l'ha sempre voluto fare e lo confermiamo oggi con il voto positivo a questo provvedimento. *(Applausi)*.

quanto sia necessario e urgente rafforzare la cybersicurezza nazionale del sistema Italia a tutti i livelli. dalla necessità di mettere in atto nuove e più concrete disposizioni - da un lato - ma anche altri strumenti - dall'altro lato - per conseguire quella elevata capacità di protezione e di risposta di fronte alle emergenze cibernetiche in forte incremento - come qualcuno ha ricordato - anche in seguito ai gravi conflitti internazionali in atto. è in gioco la sicurezza degli Stati, del nostro Stato, ma anche di settori privati di straordinario valore strategico della ricerca, della difesa e di delicatissimi apparati finanziari dello Stato. L'invasione cibernetica che un regime autoritario come quello di Putin pratica in molti modi e direzioni, come quelli denunciati ieri anche dal nostro Presidente della Repubblica, ne è una conferma. Collegata a questa c'è un'altra questione: la necessità e l'urgenza di migliorare e innovare gli apparati anche per contrastare più incisivamente la criminalità organizzata, la quale, come è noto, ha investito miliardi dei suoi proventi illeciti per criptare le proprie piattaforme evitare che esse possano essere penetrate dalle forze che contrastano la criminalità organizzata, ma anche, di contro, per aggredire e penetrare a sua volta piattaforme, comprese quelle pubbliche.

che richiedono invece la massima protezione. Nessuno può negare che ci sia un'urgenza di intervenire seriamente in questo campo. L'obiettivo che avremmo dovuto raggiungere e dovremmo raggiungere è legato quindi al conseguimento di un alto livello di cybersicurezza attraverso tutta una serie di strumenti, e soprattutto cercando di proteggere l'intero sistema del Paese,

solo nominale perché il Governo, sostenuto dalla maggioranza, ha deciso di approvare queste norme a invarianza finanziaria. In buona fede, come si può pensare di attivare queste misure per sviluppare le capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta per prevenire e gestire incidenti di sicurezza informatica, nonché attivare misure per per la prevenzione e il contrasto dei reati informatici, senza avere risorse economiche e finanziarie a disposizione? Ci saranno anche nuovi oneri e nuovi impegni per l'insieme delle amministrazioni, e non solo per lo Stato centrale, ma anche le Regioni e le città metropolitane, le Province, i Comuni, le società di trasporto pubblico e le partecipate. Oneri e impegni giusti, ma zero risorse destinate: questo la dice lunga

pur avendo nuovi oneri e nuovi impegni cui far fronte, non hanno titoli per accedere alle risorse previste dal PNRR. Anche questo rischia di essere una scatola vuota. Se poi queste amministrazioni non rispetteranno questi impegni, saranno sottoposte a sanzioni, sicuramente anche queste onerose. Insomma, si dice che la cybersicurezza ha un ruolo strategico, ma al tempo stesso, pur riconoscendo questo, non si danno, a tale settore e alle innovazioni, le gambe per camminare. Tutti i nostri emendamenti sono stati respinti, certo, con la solita, classica e ormai abituale motivazione che non ci sono risorse, della contrarietà del MEF e della Ragioneria generale dello Stato. Allora, perché

i suoi coriandoli, ma, a parte il G7, ci sono direttive europee ancora da recepire. Forse, un supplemento di attenzione il Governo e la maggioranza potevano dedicarlo. Si poteva lavorare tutti insieme, perché nessuno nasconde l'esigenza di potenziare il settore per reperire risorse ulteriori e aggiuntive, con fantasia, in interlocuzioni anche continentali. Invece, tutta questa fretta rischia di essere coperta

trovare cittadinanza. Del resto, mi permetto, semplicemente per storia, di ricordare come nel 2013 fu il Governo Monti, con la strategia

nel 2018; nel 2019, con il Governo Conte II, il perimetro della sicurezza nazionale cibernetica; infine il Governo Draghi nel 2021, con l'istituzione dell'Agenzia nazionale. Con ciò voglio dire che c'è stato un percorso che ha visto anche un coinvolgimento di tante forze

Infine, abbiamo proposto emendamenti che erano seri, assieme a quelli di tutte le altre forze delle opposizioni. Le risorse finanziarie, che non ci sono, erano contenute in emendamenti, che prevedevano anche la formazione continua del personale dedicato, la creazione di albi specialistici, l'indicazione di referenti e responsabili nelle pubbliche amministrazioni. Abbiamo proposto - come ricordava anche il senatore Bazoli nel suo intervento - quella sorta di legittima difesa nel caso di reazioni, legittime, esercitate da soggetti pubblici e privati nazionali nei confronti di intrusioni, spionaggi, hackeraggi, furti informatici; emendamenti

anche questo rischia - mi limito a questo verbo - di inserirsi in un clima nel quale a questo Governo e questa maggioranza l'indipendenza della magistratura e la separazione dei poteri danno fastidio. siamo quindi di fronte a un provvedimento bandiera, che evidenzia i problemi, dà alcune indicazioni, ma non dà a tali indicazioni, a queste normative, le gambe per camminare.

pensiamo che sia necessario (non solo giusto) lavorare insieme, anche quando il provvedimento per noi è insoddisfacente. Signora Presidente, onorevoli colleghi, viviamo senza dubbio tempi difficili e complessi. Nella massiva, inarrestabile e penetrante emersione digitale del secolo che viviamo, le potestà regolatorie di un Parlamento nazionale, ma anche delle stesse istituzioni europee, avranno nel prossimo futuro un compito particolarmente arduo. Siamo in una fase già ben più che embrionale della costituzione di veri e propri nuovi Stati digitali, particolarmente evoluti, sconosciuti nel passato, che sovvertono completamente la tradizionale natura costituzionalistica di ordinamenti basati sull'esercizio della sovranità territoriale. In questo senso gli ordinamenti statuali e anche quelli sovranazionali dovranno continuamente e repentinamente evolvere, non soltanto per preservare gli ambiti tradizionali della sicurezza e della difesa, ma le stesse economie nazionali, quando non anche gli stessi assetti istituzionali, rispetto alle minacce crescenti provenienti da mondi e universi ormai completamente iperconnessi. Addirittura a livello europeo si contrappongono già due modelli diversi: quello del costituzionalismo digitale, che prova a riproporre all'interno dello spazio cibernetico lo stesso principio liberaldemocratico della tutela degli utenti e del libero approccio alle reti, e un modello, una *policy* diversa di sovranità digitale, che punta quantomeno a preservare l'indipendenza tecnologica delle istituzioni.

delle tecnologie avanzate, più significativo e più rappresentativo della distinzione, nell'ambito dell'esercizio dell'attività di governo, tra iniziative episodiche, spesso frutto di dati emergenziali, e approccio di sistema, tra politiche di breve periodo e visione strategica. *(Applausi)*. In questo senso non vi è dubbio che il Governo presieduto da Giorgia Meloni abbia già, anche con questo provvedimento, compreso prima e dimostrato poi che il tema della cybersicurezza è divenuto questione prioritaria e strategica per la sicurezza nazionale ed a questo tema bisogna informare l'attività tutta del Parlamento. Se questo è vero in tempi di pace, lo è a maggior ragione in tempi di conflitti internazionali o di guerre ibride come quelle che stiamo vivendo, laddove vengono sistematicamente posti sotto minaccia la sicurezza informatica, quella cibernetica, quella militare e, con esse, la stessa convivenza sociale all'interno degli Stati nazionali e quindi sono messi a rischio i diritti fondamentali dei cittadini.

è finalizzato proprio a rispondere alla crescente offensiva di aggressioni al nostro ordinamento poste in essere attraverso mezzi informatici e telematici, ma in una visione più ampia tende ad ampliare il perimetro della Difesa digitale nazionale e ad apportare strumenti più efficaci, più immediati di risposta alle aggressioni in corso. Questo è, oggi, particolarmente prezioso nel rispetto della direttiva europea NIS2, con una nuova strumentazione operativa, perché è probabilmente vero che la terza guerra mondiale sarà necessariamente e inevitabilmente una guerra informatica o cibernetica, soprattutto laddove, come è stato vaticinato, la stessa intelligenza artificiale è potenzialmente più perniciosa, invasiva e pericolosa di quanto non lo siano ad oggi gli stessi armamenti nucleari. Ma un conflitto su una scala minore, subdolo e strisciante è già in atto non soltanto sullo scacchiere mondiale, ma anche nel contesto europeo e nazionale. I dati, Presidente, signori del Governo, sono particolarmente allarmanti, se consideriamo che a livello mondiale si registrano 2.200 attacchi cibernetici al giorno, con una media di un attacco ogni 39 secondi, ma il dato è allarmante anche e soprattutto per quanto riguarda lo scacchiere nazionale, non soltanto sui numeri assoluti - 1.400 attacchi all'anno, 140 al mese significa potenzialmente quattro attacchi ogni giorno - ma soprattutto perché, in percentuale, nell'ultimo periodo l'Italia è divenuta obiettivo delle aggressioni dell'11 per cento degli attacchi telematici su scala mondiale, il che non si giustifica né con riferimento al rapporto con la popolazione, né nel raffronto con il prodotto interno lordo. Dal punto di vista qualitativo, il che è ancora più inquietante, abbiamo la follia di un aumento nell'anno 2023 rispetto all'anno precedente del 27 per cento rispetto ai reati informatici legati alla criminalità ordinaria, una soglia fisiologica, e abbiamo un aumento del 625 per cento degli attacchi di matrice politica, l'80 per cento dei quali proviene proprio dal contesto geopolitico dei conflitti internazionali in corso: Ucraina e Medio Oriente. A fronte di questo scenario, Governo e Parlamento hanno non soltanto il vincolo tassativo tassativo di potenziare gli strumenti già esistenti a legislazione vigente, ma anche e soprattutto la necessità di individuare nuovi strumenti più raffinati, più efficienti, più tempestivi, che consentano una reazione adeguata. Il provvedimento va esattamente in questa direzione, perché delinea una serie di strumenti assolutamente nuovi, il primo dei quali la necessità della tempestiva segnalazione da parte di tutte le amministrazioni pubbliche rispetto agli attacchi cibernetici, perché soltanto attraverso questo sistema è possibile rendere capillare la risposta in termini di reattività e resilienza rispetto agli attacchi in corso, e poi, naturalmente, un forte inasprimento delle sanzioni penali per tutti i reati informatici. vi è l'adeguato aumento delle sanzioni amministrative, anche per i reati presupposto per la responsabilità penale delle persone giuridiche. Cito inoltre l'introduzione del reato specifico della estorsione cibernetica. Poi quel che più conta: estensione del regime delle intercettazioni previsto per la criminalità organizzata anche ai reati informatici, che vengono quindi posti sotto il coordinamento della procura nazionale antimafia, come logica desunzione, fortissimi momenti di coordinamento tra l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza e la Direzione nazionale antimafia per quanto riguarda la tutela delle infrastrutture critiche, e con le procure ordinarie per quanto riguarda la preservazione delle fonti e dei mezzi di prova. Sono inoltre previsti protocolli di sicurezza, investimenti in formazione e tecnologie avanzate. Questa è la necessità che si avverte in questo momento. con il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia, in tutta onestà, esprimo un apprezzamento sincero a tutto il Parlamento, alle forze dell'opposizione per la maturità che hanno dimostrato nel rendere possibile una celere approvazione di questo provvedimento necessario. Rivolgo un convinto plauso al Governo per la sua sensibilità su questa materia specifica, perché noi abbiamo la consapevolezza che anche in questo ambito l'Italia di Giorgia Meloni vuole svolgere un ruolo da protagonista, una grande partita di competitività e di efficienza che abbia al centro la tutela delle nostre infrastrutture informatiche pubbliche e private, la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, ma soprattutto, come sempre, la difesa dell'interesse nazionale.

testata «Fanpage» condotta all'interno di Gioventù Nazionale, l'organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia, il partito di cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è *leader* assoluta, emerge un legame diretto, reiterato ed inquietante con simbologie e parole d'ordine apertamente neofasciste. L'inchiesta mette in evidenza come Gioventù Nazionale sia organizzata su un doppio livello: un'immagine pubblica apparentemente decorosa, che nasconde in realtà condotte e prove di fedeltà e di militanza che rappresentano una continua, voluta, pianificata apologia del fascismo. Tutto ciò senza vergogna addirittura nel citare, nei colloqui tra dirigenti, il «Mein Kampf» di Hitler, che - voglio ricordarlo - è l'origine della teoria dello sterminio di ebrei, rom, omosessuali, disabili, avversari politici *(Applausi)*; e senza vergogna nel professare ammirazione per i terroristi neri dei NAR che - voglio ricordarlo - sono responsabili di lutti atroci e della strage neofascista che spezzò la vita a centinaia di persone alla stazione di Bologna la mattina del 2 agosto 1980. Presidente, tutto questo non riguarda dei "cani sciolti", ma giovani esponenti politici già in carriera, già introdotti nelle segreterie che contano, vezzeggiati da parlamentari di Fratelli d'Italia, come abbiamo visto nell'inchiesta, omaggiati pubblicamente da Giorgia Meloni come esempio di militanza. Presidente, noi vogliamo risposte sul rischio che in realtà, dietro gli elogi pubblici, dentro Gioventù Nazionale rispunti la mala pianta del fascismo, della violenza nel febbraio 2023, davanti al liceo Michelangelo di Firenze due studenti sono stati vittima di un pestaggio squadrista da parte di Azione Studentesca, che è costola di di Gioventù Nazionale. Su tutto questo non si può tacere! E invece c'è un silenzio imbarazzante dei vertici della destra, a fronte anche di provocazioni continue di candidati locali. Quelle immagini, con giovani dirigenti che inneggiano a simboli fascisti e nazisti, sono uno sfregio. Nel nostro Paese l'apologia di fascismo è un reato, voglio ricordarlo. *(Applausi)*. E sono un insulto quelle immagini! Un insulto a chi diede la vita per riscattare per riscattare il nostro Tricolore dal fascismo; un insulto a chi, "per la sola colpa di esser nato", venne condotto a morire in un campo di sterminio; un insulto a tutti i cittadini italiani, senza distinzioni. E c'è poi, Presidente, in quei video, l'ammissione di una pratica di finanziamento attraverso l'aggiramento delle norme sul servizio civile nazionale. Sono risorse pubbliche, dei contribuenti, e vogliamo chiarezza anche su questo! Oggi sarà alla Camera il ministro Piantedosi: lo ascolteremo, ma non potrà bastare. Chiediamo che venga a riferire in Aula Giorgia Meloni *(Applausi)*, che è Presidente del Consiglio e presidente di Fratelli d'Italia, di cui Gioventù Nazionale è un pezzo importante, sostenuto politicamente e finanziariamente. Chiediamo che la presidente Meloni dica cosa pensa di quei video: se è quella la militanza di Gioventù Nazionale che in pubblico ha tanto elogiato. Chiediamo che dica cosa intende fare, sulla base del giuramento che ha fatto sulla Costituzione, per debellare le forme di neofascismo, ovunque e nelle organizzazioni giovanili del suo partito. La presidente Meloni ha il dovere di parlare, per rispetto

evidenziando la sperequazione che ha visto il Mezzogiorno altamente penalizzato. Ebbene, il testo accende un faro sulle criticità connesse al Fondo di solidarietà comunale, dotazione istituita dall'articolo 1, commi da 380 a 394, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013), per ridurre il divario tra i Comuni italiani ed assicurare un'equa distribuzione delle risorse verso tutti gli enti comunali. Ecco la storia. Nel 2015 per la prima volta si applicò il Fondo di solidarietà comunale. L'ANCI e il Governo, in occasione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ridussero il tasso perequativo dal 100 per Fu previsto così che il raggiungimento del 100 per cento della perequazione dovesse avvenire nell'anno 2021, ma tale previsione è stata successivamente sospesa. Mi chiedo perché. Ecco la risposta: è sicuramente una strategia politica e/o dei veri artifici tecnici per trasferire risorse dal Sud al Nord. Così ad oggi, in luogo della perequazione integrale, la quota di risorse raggiunge appena il 52,5 per cento e il completamento della transizione è previsto - udite, udite - solo per il 2030. Ebbene, come riporta il libro «Zero al Sud», l'ex presidente della Commissione bicamerale sul federalismo, il ministro Giorgetti, cercò di capire se, anziché il 45,8 per cento, si potesse usare il criterio del 100 I dati - disse il Ministro in audizione - sarebbero scioccanti; magari ce li facessero avere in modo riservato, o in una seduta segreta, come avviene in Commissione antimafia. Sì, avete capito bene: sin dal 2015 i territori fragili hanno ricevuto una perequazione dimezzata, cioè l'esatta metà di quanto dovrebbe essere garantito ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione. Si è deciso di secretare i dati, proprio come si fa in Commissione antimafia. Onorevoli colleghi, la novità è che finalmente abbiamo i dati completi. La settimana scorsa, infatti, il presidente, dottor Arachi dell'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) è intervenuto nel corso di un'audizione parlamentare sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale, portando alla nostra attenzione diverse tabelle, calcoli e passaggi altamente tecnici, dove, in uno stralcio, si può per la prima volta in assoluto certificare lo scippo che il Mezzogiorno ha subìto a seguito della mancata applicazione della perequazione integrale del Fondo di solidarietà comunale. Come si legge a pagina 30 di una memoria depositata dall'Ufficio parlamentare di bilancio in Commissione, «la mancata applicazione integrale applicazione integrale dei criteri *standard*, penalizza in media significativamente il Sud, per 31,9 euro *pro capite* (…), mentre favorisce il Nord-Ovest, per 17,2 euro *pro capite*, e soprattutto il Nord-Est, per circa 23,3 euro *pro-capite*». Effettuando un calcolo basato sulla popolazione residente delle macroaree, ho così appreso che lo Stato ha privato il Mezzogiorno di 638 milioni all'anno e cioè oltre 5 miliardi dal 2015, drenando al Nord maggiori risorse per oltre 4,4 miliardi, come certificato dall'UPB il 29 maggio 2024. Inoltre, la cosa grave è che questo Governo, dopo aver depennato i 16 miliardi di risorse destinate al Sud dal PNRR, sottratto ai Comuni fragili diversi miliardi dal Fondo di solidarietà comunale (FSC) e sforbiciato quattro miliardi dal Fondo perequativo infrastrutturale destinato al Meridione, ha poi fatto sì che fosse approvato questa mattina - e tutti lo sapete lo sapete - in seconda lettura l'autonomia differenziata, che spaccherà l'Italia in due. Pertanto, compito dell'opposizione è vigilare sull'assegnazione dei fondi FSC e PNRR e denunciare il furto che questo Governo sta attuando ai danni del popolo meridionale.

delle imprese e del *made in Italy* (mi pare si chiami così adesso il Ministero dello sviluppo economico) a rispondere a un'interrogazione che ho posto al Ministro il 25 gennaio - quindi, andiamo a festeggiare i sei mesi da quel giorno

dei passi più importanti fatti finora verso la creazione di un sistema che riunisca tutto il mondo del tessile, dell'accessorio, della pelle e quant'altro. Confindustria moda è nata e poi inopinatamente si è sciolta, perché un pezzo grosso, Sistema moda Italia, la parte del tessile, ne è uscita e altri pezzi si stanno perdendo per strada. Ho chiesto al ministro Urso di farmi sapere se sia al corrente di questa cosa e cosa ne pensi. Parliamo tanto di fare sistema e quando poi il sistema si sgretola, il Governo probabilmente neanche se ne accorge. La cosa grave è che io gli ho chiesto sei mesi fa di questo problema e non ho avuto alcuna risposta. Credo che il Governo sia proprio tenuto a rispondere agli atti di sindacato ispettivo, al Parlamento che gli dà la fiducia. Credo sia intollerabile far attendere sei mesi un parlamentare, anche perché poi le situazioni evolvono, quindi, se il Governo non ne era al corrente a gennaio e ancora non mi risponde, mi verrebbe da aggiungere un ulteriore interrogativo: cos'è successo tra gennaio e giugno? La pregherei

Ricordo che martedì 25 giugno, alle ore 12,30, è convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Voteranno per primi gli onorevoli senatori. **Sui lavori